Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché del parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto a seguito della scomparsa della senatrice Cecilia Donaggio, ha riscontrato, nella seduta odierna, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista alla quale apparteneva la predetta senatrice è Sandro Spinello. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Sandro Spinello. Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di 20 giorni per la presentazione di eventuali reclami. Onorevoli colleghi, lo scorso 30 dicembre tutto il mondo ha appreso con commozione che la senatrice Rita Levi-Montalcini aveva concluso, alla veneranda età di 103 anni, la sua straordinaria esistenza terrena. Insigne figura di donna e di scienziata, il suo rilevantissimo contributo al progresso delle scienze neurologiche, che le valse il premio Nobel per la medicina nel 1986, non esaurisce la multiforme ricchezza del suo eccezionale profilo. Le tappe fondamentali della sua carriera scientifica sono universalmente note. In primo luogo, la laurea in medicina e chirurgia a Torino, nel 1936, conquistata con determinazione e volontà in un contesto familiare e sociale poco favorevole all'impegno femminile in campo scientifico. Poi l'emigrazione in Belgio, con il suo maestro Giuseppe Levi, per sfuggire all'infamia delle leggi razziali. I fortunosi studi nel periodo bellico, il trasferimento negli Stati Uniti, dove la ricerca visse i primi sviluppi fondamentali che portarono alla decisiva scoperta del fattore di accrescimento della fibra nervosa. Seguirono poi il ritorno in Italia nel 1977, con i prestigiosi incarichi di direzione e di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche, fino al conseguimento del premio Nobel per la medicina nel 1986. Membro di alcune tra le più importanti istituzioni culturali internazionali, con la sua profonda passione ha alimentato negli anni una instancabile attività di promozione della ricerca e della cultura scientifica, rivolta in particolare alle giovani generazioni, in linea con quello spirito di generosa condivisione del proprio sapere che l'aveva portata a contribuire allo sviluppo di centri e linee di ricerca che sono ancora oggi all'avanguardia nel mondo. In quest'ottica si sviluppa sia l'azione della Fondazione Levi-Montalcini, orientata all'assistenza dei giovani nella scelta del percorso di studio e di lavoro ed alla valorizzazione del contributo femminile al progresso della società, sia l'attività scientifica dell'Istituto europeo di ricerca sul cervello, fondato nel 2005. Nel settembre del 2001 Rita Levi-Montalcini entrò a far parte nella nostra Assemblea, nominata dal presidente Ciampi senatrice a vita per altissimi meriti in campo scientifico e sociale. La sua figura illustre ha sempre costituito un'alta testimonianza delle conquiste del genio italiano nel mondo ed, insieme, un monito a continuare ad investire energie e fondi nella ricerca scientifica, in particolare in quella direttamente rivolta a comprendere i meccanismi di funzionamento del nostro corpo e della nostra mente e a combattere le malattie più gravi. Come scrisse Primo Levi nel 1986, all'indomani del conferimento del premio Nobel, in Rita Levi-Montalcini convivevano una volontà indomita e un piglio principesco, accanto a quella rara combinazione di pazienza ed impazienza che è propria di grandi innovatori: tutte qualità necessarie ad infrangere la barriera dell'ignoto e ad avvicinare l'umanità alla meta più evanescente e gelosa, quella della mente umana che comprende se stessa. È allora in questo spirito di commossa riconoscenza che esprimo, a nome di tutta l'Assemblea, la vicinanza del Senato ai familiari e ai collaboratori di Rita Levi-Montalcini e invito tutti i colleghi a onorare la sua illustre memoria osservando un minuto di silenzio e di raccoglimento.

Onorevoli colleghi, come purtroppo è tristemente noto,

ed aveva continuato come studentessa lavoratrice a coltivare la sua formazione fino a laurearsi in scienze politiche all'università di Padova nel 1974. L'acuta passione politica e lo spiccato senso di giustizia sociale la spinsero da subito ad impegnarsi per la difesa dei diritti dei lavoratori. L'attività sindacale in seno alla CGIL condurrà Franca Donaggio a ricoprire incarichi di responsabilità, da segretario provinciale e regionale della Federazione dei lavoratori del settore energia a coordinatrice delle donne della CGIL e a presidente del comitato delle donne della Confederazione europea dei sindacati. Nel maggio 2006, in occasione della formazione del secondo Governo Prodi, Franca Donaggio fu nominata Sottosegretario di Stato per la solidarietà sociale. Eletta senatrice nella Regione Veneto al principio della XVI legislatura, entrò a far parte di questa Assemblea nella quale fu componente attiva e autorevole della Commissione permanente lavori pubblici, comunicazioni e segretario della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle morti bianche. Nonostante il terribile incedere della malattia, affrontata con il coraggio e la determinazione tipici della sua tempra forte e instancabile, tutti noi ricordiamo il suo contributo di impegno e di passione dedicato fino all'ultimo a sostegno della coesione sociale e dei diritti dei più deboli. Nel manifestare la vicinanza del Senato ai familiari, agli elettori di Franca Donaggio e ai colleghi del Gruppo parlamentare del Partito Democratico, invito l'Assemblea ad osservare un munito di silenzio e di raccoglimento nella memoria commossa della nostra collega, il cui rientro ricordo perfettamente e che avevamo salutato tempo or sono. sono. Raggiungendomi ai banchi di questa Presidenza per ringraziarmi, nell'abbracciarmi aveva ribadito di essere una grande lottatrice. Mi disse: io sono una grande lottatrice e continuerò a combattere. L'abbracciai con più affetto e le dissi: combatti, siamo tutti con te. Rimarrà con noi.

signora Presidente, colleghi senatori Ricordiamo oggi una donna che, con la sua lunga esistenza, ha attraversato la storia, ha onorato la scienza, ha onorato signor Presidente. Ricordiamo oggi una donna che, con la sua lunga esistenza, ha attraversato la storia, ha onorato la scienza, ha onorato il nostro Paese nel mondo, ha onorato l'umanità e, per oltre dieci anni, ha onorato anche questo Senato della Repubblica. Il secolo abbondante trascorso su questa terra da Rita Levi-Montalcini non ci lascia solo la scoperta dell'NGF, il fattore di crescita nervoso che le valse il premio Nobel e che tante prospettive ha dischiuso per la speranza di cura di malattie gravissime. Ci lascia anche un insegnamento di vita scolpito nella sua attività di scienziata, ma anche nel suo impegno sociale e nelle tante testimonianze che, attraverso i suoi libri, ha dedicato soprattutto ai più giovani. Ci lascia una grande scuola, diffusa su tutto il territorio nazionale, impegnata ad approfondire quella scoperta che dopo sessant'anni rappresenta ancora una novità, presenta tutt'oggi molte potenzialità per il bene dell'umanità e racchiude in sé le radici della cura di molti mali pesanti. Dell'uomo, Rita Levi-Montalcini amava soprattutto l'imperfezione. Come nell'errore risiede la scintilla dello sviluppo scientifico e intellettuale, così nel suo essere imperfetta risiede la meraviglia dell'umanità e la sua capacità di evolversi. Per questo ella, che ha conosciuto gli orrori del Novecento, non ha mai perso fiducia nel desiderio dell'uomo di conoscere, in quella spinta a continuare a cercare che è poi motore del progresso scientifico. Ai giovani raccomandava impegno e senso di responsabilità, che riteneva motivo dei suoi risultati ancor più dell'intelligenza che, nonostante il suo schermirsi, noi sappiamo essere stata straordinaria. Si è molto spesa per la partecipazione delle donne alla vita pubblica in diverse latitudini del mondo, affermando le pari capacità, lottando per le pari opportunità, ma anche valorizzando le differenze come una ricchezza da non annullare. E malgrado non vivesse una dimensione religiosa, coltivava un profondo senso etico, dell'onore, dell'impegno, del rispetto e della responsabilità verso gli altri. Lo dico, signor Presidente, pur non avendo sempre condiviso alcune sue riflessioni, ad esempio sulla fine della vita. Della scienza nutriva una concezione umanistica, di impresa di conoscenza al servizio della dignità dell'uomo. Una concezione che, come ha ricordato il professor Giorgio Israel nei giorni della sua scomparsa, le aveva fatto definire ripugnanti alcune ricerche sulla clonazione. Una concezione che l'aveva portata a non unirsi mai al coro di chi considera oscurantista qualsiasi obiezione a qualsiasi sviluppo della ricerca, e a criticare applicazioni che riteneva incompatibili con i principi di un'etica umanistica. Rita Levi-Montalcini rifiutava le visioni totalitarie: per lei il concetto di verità assoluta non rientra tra le finalità della scienza, che è soddisfazione del desidero perenne di perenne di conoscere posto al servizio dell'umanità. Della scienza ella aveva una visione complessiva. Riteneva che non potesse ridursi a un'analisi dei percentili: sarebbe stato come contemplare un mosaico soffermandosi sulle singole tessere senza cogliere il disegno d'insieme. La scienza, per lei, è in grado di rispondere alle richieste del nostro tempo solo se non si perde di vista il bisogno di conoscere la globalità dei fenomeni. La chiave del suo straordinario percorso esistenziale, insomma, risiede nell'uomo. Anche nella curiosità che nutriva per le nuove tecnologie, la sua attenzione era rivolta soprattutto ai "nuovi Magellani" (così li definiva), giovani navigatori nell'era della modernità. Proprio ai giovani Rita Levi-Montalcini lascia la sua eredità più preziosa, perché la scienza sia al servizio del bene comune e gli strumenti della tecnologia vengano impiegati per combattere le piaghe anche sociali del nostro tempo: l'analfabetismo, il razzismo, quella povertà che tanto l'aveva emozionata a Rio de Janeiro, la notte di Capodanno di sessant'anni fa, nei giorni in cui la sua intuizione trovava conferma in sede sperimentale, quando vide migliaia di "senza casta" scendere in spiaggia dalle loro capanne e gettare mazzi di fiori fra le onde. È questa l'immagine che vogliamo conservare, per ricordare così, nella sua scienza e nella sua umanità, il suo contributo; ed è con questa immagine che il Gruppo del Popolo della Libertà le rende omaggio.

Credo che bisognerebbe riflettere un po' anche sul fatto che l'esperienza scientifica di Rita Levi-Montalcini esprime un modo di intendere la stessa funzione della scienza e la stessa funzione dello scienziato non come individualità (lo scienziato) e neanche come fatto isolato, vicenda personale (il percorso scientifico), ma al contrario lo scienziato come soggetto che agisce in un percorso in relazione con altri per uno scopo esterno che non la propria ambizione o la Grazie Grazie per il fatto di essere riuscita a creare in breve tempo un gruppo di ricercatori americani, tra cui moltissime giovani donne che - mi diceva - sono più brave dei ragazzi. Questo già descrive la personalità di Rita Levi-Montalcini, che si ritrova con le stesse caratteristiche negli altri ambiti del suo impegno: quello sui temi sociali e sui temi civili. Molti hanno ricordato la Fondazione la Fondazione Rita Levi-Montalcini, di cui ho l'onore di essere componente nel consiglio d'amministrazione al posto di Tullia Zevi, una fondazione orientata al progresso culturale e scientifico di giovani donne africane. africane. Il suo impegno in questo campo partiva dalla consapevolezza che ogni limite allo sviluppo nei Paesi che questo limite registrano nel mondo trova nel protagonismo delle donne la sua prima inarrestabile forza di superamento. Non era quindi soltanto un solidarismo compassionevole, come taluno un po' superficialmente talvolta lo ha descritto, ma, al contrario, un contributo vero che Rita intendeva dare con la sua fondazione e che la fondazione continuerà a dare con il suo lavoro nel ricordo di Rita: un contributo all'emancipazione e al progresso di tanti Paesi del mondo attraverso l'emancipazione e il progresso, tramite il suo sapere, di tante donne del mondo.

il suo compiacimento, venato anche da una certa ironia, quando mi raccontava di quanto era diventata brava a preparare documenti falsi: «Sai, noi scienziati siamo bravissimi in questa opera di fino». I suoi libri e l'attività che svolse nella scuola, anche nel momento in cui diventò presidente dell'Enciclopedia Italiana, avevano questo scopo, che era appunto altro da sé: una promozione del sapere e, insieme, una promozione delle volontà. È questo il senso del libro «Senz'olio contro vento», che tra i primi Rita Levi-Montalcini consegnò alle stampe: un inno alle capacità dell'uomo e

tramandava, o meglio, raccontava ai giovani, senza mai assumere come archetipo e modello la propria vita, ma con questa capacità di comunicazione di esperienza, insieme alla forza della sua Potremmo dire che era sorretta da una grande fede illuministica, fondata sul primato della razionalità, ma insieme da una profonda fede umanistica, celebrata nella fiducia e nella capacità umana di svilupparsi, di crescere e di resistere nella difficoltà. Aveva questa abilità di esercitare una funzione pedagogica senza pedagogia, mettendo sempre - come dicevo prima - la propria esistenza a dimostrazione, non a modello, di come possa essere fatto. Qualcuno ha ricordato in questi giorni una frase che

Mi ha colpito, come credo abbia colpito tutti, il fatto che dall'emanazione delle leggi razziali e dalle limitazioni che conseguentemente le vennero allo studio e alla ricerca seppe trarre grande forza. La prima volta che la conobbi, le sentii dire una cosa che sul momento mi colpì moltissimo, e che invece le ho sentito dire più volte e ho trovato poi congeniale al suo modo di essere, quindi non più sorprendente:

Questo voglio dire quando racconto del fatto che sapeva essere pedagogica senza pedagogia e sapeva mettere in guardia dalla paura, invitando sempre al coraggio, anche quando l'ostacolo sembra insormontabile. Anche il suo impegno sul carcere, che molti conoscono e che ho avuto il piacere di condividere, era segnato dalla stessa volontà di introdurre gli elementi della razionalità e del progresso in un campo troppe volte segnato da un intervento che si muove sul filo talvolta anche un poco ipocrita della compassione. Rita voleva soltanto dare un'occasione, un'occasione ancora alle donne che stavano

Torino, anche se ciò è stato spesso letto come vanità, mentre avvertiva il dovere nei confronti di se stessa e degli altri di dare un'idea dignitosa di Tutto questo non le toglieva quella amabilità e quella capacità di entrare in relazione simpatica con il mondo, in una relazione che era asciutta, ma sempre seria, impegnativa e profonda.

È una presenza alla quale ci lega un grande affetto. Arrivò qui in Senato come senatrice a vita, nominata, appunto, dal presidente Ciampi. Chi l'ha conosciuta in quest'Aula ha avuto due scelte, entrambe, devo dire, praticate: quella di profittare del privilegio di conoscerla, di conversare con lei, di osservarla e di ascoltarla; oppure quella di disprezzarla, con termini e con toni di efficace bassezza, senza riservarle neanche quella degnazione ipocrita che pure si usa in quest'Aula nei confronti degli avversari che non si stimano. Questo ovviamente non ha tolto niente a Rita Levi-Montalcini. Io credo che, invece, continui a togliere a coloro che lo fecero, perché è mia opinione che era comunque lei, qui, con i suoi 40 chili scarsi, gli occhi che più non vedevano, con il suo bastone, la fragile prova dell'umana grandezza.

ampiamente illustrato tutti i meriti in campo scientifico e in campo pubblico e tutte le tappe della carriera, anche accademica, della professoressa Rita Levi-Montalcini, della senatrice a vita Rita Levi-Montalcini. le parole dei colleghi che mi hanno preceduto sono state toccanti e hanno messo in evidenza l'importanza e la rilevanza di questa figura non solo scientifica, ma direi pubblica nel nostro panorama culturale, scientifico e politico. Scompare una delle menti più lucide ed eccelse. Il Gruppo della Lega Nord rivolge un sentimento di vicinanza ai parenti e ai collaboratori della senatrice a vita Rita Levi-Montalcini. Il 1° agosto del 2001 il presidente Ciampi la nominò senatrice a vita per aver illustrato la nostra Repubblica con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale,

scientifica: «La mancanza di complessi, una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta e la noncuranza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti (...), mi hanno enormemente aiutato a far fronte agli anni difficili della mia vita». Credo che in queste parole siano ben evidenti la determinazione e il coraggio di una donna che, pur in un momento non facile per il genere femminile (stiamo parlando dei primi anni del ventesimo ce la mise tutta, con impegno, per fare carriera nel mondo scientifico e poi rivestire un ruolo così importante nel mondo pubblico e anche in quest'Aula, che

un'altra persona grandissima, Primo Levi, definì la senatrice Rita Levi-Montalcini: «una piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa». Credo che in queste poche parole sia condensato il senso della nostra riconoscenza come Gruppo della Lega Nord. Signora Presidente, onorevoli colleghi, è per me un onore oggi intervenire in occasione della commemorazione della senatrice Rita Levi-Montalcini. Sebbene ogni parola potrebbe apparire superflua di fronte ad una tale elevata personalità, non posso qui che ricordare, con immensa stima, una delle donne che maggiormente ha rappresentato il nostro Paese in settori fondamentali come quello della ricerca e delle scienze sociali. Ma non solo. Il riconoscimento a Rita Levi-Montalcini, infatti, va oltre. Nonostante la sua vita sia stata pienamente dedicata allo studio nel settore della medicina, ad essa va riconosciuto il merito di non essersi mai sottratta ad impegni e lotte civili che riteneva fossero fondamentali al Paese. Era una donna moderna, nonostante l'età e nonostante abbia vissuto l'intero arco del secolo scorso vivendo sulla propria pelle le vicissitudini storiche che noi tutti conosciamo. Ha affrontato le due guerre mondiali conoscendo in prima persona le conseguenze delle leggi razziali e l'obbligo di lasciare la propria patria per un'appartenenza etnica allora inaccettabile. Tutto questo, senza mai interrompere i suoi studi, senza mai arrendersi e raggiungendo con estremo impegno risultati ambiziosissimi. Con la stessa tenacia, mai smise di proporre, assecondare ed avallare le battaglie civili e sociali che riteneva indiscutibili. Anche sottoponendosi a critiche politiche che per la sua prioritaria natura scientifica non le spettavano. Ritengo oggi che una donna come lei non possa che essere da esempio in una società che lentamente declina. La sua forza, il suo impegno e anche il suo orgoglio - qualità che ha sempre difeso e che le ha consentito di divenire la persona che è stata - sono fuori discussione. Sempre ha insistito sull'importanza di un impegno intellettuale da parte di tutti noi; sulla necessità di ritagliare nelle vite di tutti un proprio spazio in cui mettersi in gioco e in cui evidenziare le proprie capacità e le proprie attitudini. Una donna vulcanica che molto spesso ha lasciato qualcuno di noi a bocca aperta. Qualcuno di noi che mai si sarebbe aspettato che una donna così delicata e fisicamente minuta potesse avere quella forza nelle parole e nelle battaglie per i diritti civili che resteranno impresse nella nostra storia. Oggi, in un contesto sociale e politico altamente precario, la voglio ricordare con sincera stima e personale affetto, auspicando che siano personalità come la sua ad essere un faro per tutti noi. Un esempio da cui trarre i migliori tratti e la più vera onestà intellettuale ed umana.

quanto piuttosto per l'essere stata un esempio di vita, di impegno e di correttezza. Ricordarla come colei che ha vinto il premio Nobel per la medicina è riduttivo. Ella seppe sfidare le convenzioni del suo tempo e attraversarne le mille difficoltà senza turbamento, tanto da dire: «Le leggi razziali del 1938 si sono rivelate la mia fortuna, perché mi hanno obbligata a costruirmi un laboratorio in camera da letto, dove ho cominciato le ricerche che mi hanno in seguito portato alla scoperta del fattore di accrescimento della fibra nervosa». Per sua stessa ammissione le difficoltà se le scrollava di dosso. La professoressa ci ha lasciato come messaggio, come le piaceva ricordare, non tanto quello scientifico, quanto quello di affrontare la vita con totale disinteresse alla propria persona e con la massima attenzione verso il mondo che l'ha circondata, sia quello inanimato che quello vivente. Questo, secondo lei stessa, era il suo maggiore merito. «L'unico ideale per cui abbia lavorato è stato quello di aiutare gli altri e forse per questo» - diceva - «la ricerca mi ha dato molto di più di quanto potessi sperare». Con questo atteggiamento si rivolgeva ai giovani. Ha sempre augurato loro di avere la sua stessa fortuna: quella che l'ha condotta a disinteressarsi della sua persona, ma che l'ha spinta ad avere sempre una grande attenzione nei confronti di tutto ciò che la circondava; a tutto quanto il mondo della scienza, senza trascurare i valori della società, le presentava. Come non condividere la sua convinzione secondo la quale il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori della vita? «La vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori» - diceva - «perché questi rimangono anche dopo la nostra morte». Quei valori da lei strenuamente difesi e testimoniati, tra i quali la parità di genere, e lei ne è sempre stata un esempio luminoso.

rimase ancorata alla sua lucidissima mente: «Il corpo faccia quello che vuole, io non sono il corpo, io sono la mente». Una donna, quindi, proiettata costantemente verso il futuro e particolarmente verso i giovani, a cui si rivolgeva costantemente spronandoli: «Non pensate a voi stessi, pensate agli altri». Quello che deve premerci ora, oltre ad alimentare il ricordo di questa grande italiana come esempio per le giovani generazioni, è di non disperdere il suo messaggio, il suo lavoro. Questo è quanto concretamente possiamo e dobbiamo fare, anche se non sarà sufficiente per contraccambiare quello che lei ha dato al nostro Paese, valore incommensurabile. Ma servirà a sentirla ancora viva, rispettando la sua convinzione secondo la quale: muore il corpo sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato». Alimentiamo quindi quanto lei ha fatto e ricordiamo questo suo messaggio.

dare ed ottenere un riconoscimento straordinario della condizione femminile, ebbene, pure nel dolore

Prima di rivolgermi con il pensiero e le parole alla senatrice Rita Levi-Montalcini, mi permetterà, signora Presidente, di premettere

che non ha l'ha mai lasciata e che ha voluto donare ai suoi colleghi senatori che sapevamo della sua condizione, perché non la nascondeva, e che e che vedevano la sua passione bruciare più forte del male. Credo che associare queste due donne nella commemorazione di oggi sia il più grande tributo che si possa portare alla dignità della condizione femminile nella vita pubblica e civile, oltre che nel Parlamento. La senatrice Rita Levi-Montalcini, cui mi legava personalmente un rapporto di fraternità e di devozione - se posso usare questa espressione in senso civile - ha vissuto una esistenza ineguagliabile. Rita Levi-Montalcini ha insegnato a molti che il cervello si rigenera. Ma tutto sommato ha insegnato a tutti noi che l'esercizio della conoscenza assicura il rinnovarsi e non solo il protrarsi dell'esistenza. Rita era una donna di ferro nella sua sottigliezza fisica. Non vedeva, negli ultimi anni della sua vita, ma leggeva dentro il senso delle cose come una ragazzina. Rita Levi-Montalcini aveva un inestinguibile amore per le libertà, che certo le derivava dall'appartenenza alla comunità ebraica, dalla sofferenza per le leggi razziali e dalla battaglia incessante che ha condotto per le libertà civili e democratiche. Di lei va ricordato anche l'autentico rispetto per il fattore religioso, e per ogni convincimento religioso, nella cornice inalienabile della laicità dello Stato. Ciò che Rita Levi-Montalcini ha fatto ed ha simboleggiato per la ricerca e il sapere in Italia, ciò che essa ha fatto in quanto donna, in quanto cittadina italiana, europea e del mondo

rimarrà per sempre. Voglio anche ricordare di Rita Levi-Montalcini la dimensione politica. Lei ha partecipato come senatrice a vita: spesso si dibatte sul senso della funzione dei senatori a vita, ma io voglio ricordare che nella tenace sua partecipazione, anche ad alcuni voti di fiducia nella passata legislatura, c'era uno degli elementi della coerenza del suo operato di donna, e di donna anche politica, come il riconoscimento della carica di le aveva attribuito quale funzione, nell'interesse generale che esercitava secondo i propri convincimenti. l'onore che mi ha fatto e ci ha fatto la senatrice Levi-Montalcini nel sottoscrivere, tra gli ultimi atti della sua vita parlamentare, alcuni documenti che io stesso ho presentato e che l'Assemblea del Senato ha approvato: ricordo quello del 2010 sui cambiamenti climatici e la sicurezza energetica precedentemente, quello riguardante il contrasto alla corruzione. Rita Levi-Montalcini, scienziata, donna, combattente per la libertà, figura di straordinario equilibrio politico e personale e di straordinaria dignità civile, oggi merita di essere ricordata, assieme ai suoi collaboratori. A questi ultimi va la fiducia l'apprezzamento per la generosità del lavoro svolto accanto a lei, spesso con fatica e con grande dedizione, sempre con grande apertura culturale, scientifica e civile:

che hanno dato molto, nella diversità delle loro esperienze. C'è una grande dignità nella seduta odierna del Senato. Spero, signora Presidente, che il futuro Presidente della Repubblica ricordi che le donne senatrici a vita sono state una minoranza estrema nel corso della vicenda costituzionale e repubblicana, ma forse meritano di essere più numerose. Infatti, vi sono molte donne accanto agli uomini che avrebbero meritato di essere senatrici a vita e forse nella prossima legislatura il futuro Presidente della Repubblica potrà prendere l'esempio luminoso di Rita Levi-Montalcini per proseguire su questa strada dando, non nell'equilibrio aritmetico ma in quello politico, sociale e rappresentativo, riconoscimento

Signora Presidente, ricordiamo oggi la grande figura di Rita Levi-Montalcini. Mi piace ricordarla partendo da una sua frase, una delle tante: «L'umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da entrambi i sessi». Questo diceva Rita Levi-Montalcini, che sicuramente ha rappresentato l'esempio della donna libera, come ella si sentiva. Cresciuta in un mondo dove dominava la figura maschile (eravamo agli inizi del Novecento), pur avendo come donna la stessa capacità mentale dell'uomo, l'approccio era diverso e era diverso e pertanto la donna aveva poche possibilità di emergere. Ecco perché Rita Levi-Montalcini fece la scelta di vivere senza un marito, rinunciando alla famiglia, per dedicarsi completamente alla scienza e alla neurobiologia.

Grande è stato anche il suo impegno sociale. È stata parte attiva in tante campagne di interesse politico, come quella contro le mine antiuomo, o per la responsabilità degli scienziati stessi nei confronti della della società. Sicuramente è stata una grande donna, una scienziata illuminata e un politico attento. Grande è il mio personale

non solo da ammirare, ma da seguire, perché ha dimostrato in tutta la sua vita con il suo impegno non solo grande intuizione scientifica ed intelligenza, ma soprattutto quello di cui necessita la ricerca scientifica, e cioè grande amore per la medicina.

Signora Presidente, il secolo lungo di Rita Levi-Montalcini è certamente una traiettoria esemplare sotto molti aspetti. Già i colleghi si sono intrattenuti su molti dei caratteri biografici di questa esperienza. fondativa dell'attività di ricerca degli scienziati che si muovono tra solitudine e collettività. Ma più in particolare vorrei ricordare che gli inizi dell'attività di ricerca di questa scienziata così speciale sono la fotografia di unità della ricerca scientifica che ha qualcosa di strano e di commovente; la ricerca fatta con mezzi artigianali, in rifugi di fortuna anche durante il periodo delle persecuzioni razziali, in piccolissimi laboratori allestiti con mezzi casuali; la volontà ferrea di condurre delle sperimentazioni in condizioni ambientali disagiate. Questa è un'esperienza che oggi sarebbe impossibile, che si confronta con un apparato di strutture di ricerca necessariamente costoso e complicato. - la solitudine del ricercatore e nello stesso tempo l'appartenenza a una collettività. Il premio Nobel premia un'attività eccezionale, ma ogni scienziato, ogni ricercatore sa che il suo lavoro è un piccolissimo passo dentro un cammino di conoscenza collettivo. È impossibile pensare ad un prosieguo, ad una invenzione, ad un atto creativo nell'attività di ricerca, senza che questo si fondi su una complicata messe di esperienze, una ricchissima bibliografia, rapporti internazionali, suggestioni di scuola. Questa è in un certo senso la perfetta bellezza del lavoro del ricercatore: sapere di poter dare un contributo creativo che fa scattare in là il cammino della conoscenza e nello stesso tempo sapere benissimo di essere avvolto dentro una comunità che non è presente, che è lontana e che purtuttavia imprime seduzioni, fascino, curiosità. L'altro elemento, l'altra antinomia che può essere ricordata è quella che fa riferimento ad una espressione di un altro premio Nobel, un grande genetista: il caso e la necessità. Nel lavoro dello scienziato c'è il caso, talvolta come punto di nascita dell'attività di ricerca, una curiosità che si appunta su elementi che in sé a qualsiasi altra mente non farebbero scattare nessuna fantasia e che invece nella mente del singolo creatore costruttivo di ricerca fanno inesplicabilmente scattare un meccanismo di curiosità irresistibile. Il caso. Però, nello stesso tempo, una volta approdati al momento e al tema della ricerca si imprime la potenza della necessità, la capacità di regolarsi e di regolare il lavoro sulla base delle leggi - chiamiamole così - della necessità scientifica. Molte cose ci lascia questo personaggio straordinario. Però ne voglio privilegiare una su tutte le altre: la lotta per la conoscenza e i doveri che la lotta per la conoscenza imprime a tutti noi. Noi oggi sappiamo che la ricerca scientifica non può essere affidata solo a mezzi artigianali. L'autorità politica, le assemblee elettive di un Paese hanno il dovere di rispettare in senso fondativo la necessità della lotta alla conoscenza e fornire di mezzi, risorse e strumenti tecnici, di ricchezza finanziaria. La cosa fondamentale che il Senato può fare per rispettare la memoria di Rita Levi-Montalcini è produrre uno sforzo rinnovato e potentissimo per finanziare la formazione e la ricerca e l'incoraggiamento all'ingegno, che è l'elemento fondamentale. Non possiamo lasciare gli ingegni disponibili nel mondo senza mezzi e senza possibilità di accedere alla loro materia di ricerca.

il pensiero mio e del mio Gruppo, commosso e riconoscente, va alla grande figura di una senatrice fuori dal comune, Rita Levi-Montalcini, che tanto ha rappresentato per la causa della scienza, l'affermazione delle donne, della libertà e della democrazia. Nel 1986 vinse il premio Nobel per la medicina grazie alla scoperta e all'identificazione del fattore di accrescimento della fibra nervosa. È stata, inoltre, la prima donna a essere ammessa alla Pontificia accademia delle scienze. Nel 2001, fu nominata senatrice a vita, dall'allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che la scelse proprio per i suoi meriti sociali e scientifici. È stata, come ricordava chi mi ha preceduto, una delle poche

un grande vuoto, non solo per quest'Aula, ma soprattutto per il nostro Paese, fucina di giovani talenti. Ed è a loro che mi rivolgo quest'oggi, perché possano sempre mantenere vivo nelle loro menti il ricordo e soprattutto l'esempio di una grande scienziata, di una grande donna, una figura italiana nella quale rintracciare un esempio positivo. E sul suo esempio spero che i giovani ricercatori, e in particolare - concedetemelo - le giovani scienziate, anche quelle che hanno già dato prove straordinarie in centri di ricerca europei, come il CERN di Ginevra o l'ESTEC dell'Aja, o con scarsi mezzi e molte difficoltà negli istituti di ricerca nazionali, possano proseguire il loro percorso professionale tutto in salita, conseguendo grandi successi, come ha fatto Rita Levi-Montalcini, che proprio rivolgendosi ai giovani disse: «Ai giovani auguro la stessa fortuna che mi ha condotto a disinteressarmi della mia persona ma ad avere sempre una grande attenzione nei confronti di tutto ciò che mi circonda, a tutto quanto il mondo della scienza, senza trascurare i valori della societàۚ». «Il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. Non ha importanza che siano religiosi oppure laici. I giovani devono credere in qualcosa di positivo, perché la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori, perché questi rimangono anche dopo la nostra morte. Quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato». Il Gruppo Fratelli d'Italia condivide questi principi e rende omaggio a una grande donna che ha reso fiere tutte le donne e tutto il popolo italiano.

*(PdL)*. Signora Presidente, nel corso dell'intera legislatura, Cecilia Donaggio è stata una delle colleghe più presenti, più attive e più capaci nei lavori dell'8a Commissione. In molte occasioni ha saputo fornire un contributo di qualità sui temi più complessi, dalla sicurezza dei cantieri di lavoro al trasporto, al trasporto pubblico, alla riforma dei porti. solida preparazione politica, frutto certo di un'esperienza non comune vissuta all'interno del sindacato CGIL. È stata, come ha ricordato il nostro Presidente, segretaria provinciale della CGIL a Venezia segretaria regionale del Veneto; dal 1996 al 2003, ha fatto parte della segreteria nazionale della FILT-CGIL. La scuola del sindacato le aveva sviluppato quella sensibilità non comune che l'ha portata ad essere sempre attenta al mondo del volontariato, ai temi della solidarietà, cioè al prossimo. La sua partecipazione in qualità di Sottosegretario al Governo Prodi, nel 2006, con delega alla solidarietà sociale, è stata l'occasione per dare il meglio di sé. Ricordiamo infatti l'ottimo lavoro svolto che Franca fece proprio in una delle trincee più complesse e delicate: le politiche per gli anziani, anziani, a favore dei disabili e dei disoccupati, cioè sui temi della coesione sociale. Si deve alla sua capacità e al suo particolarissimo impegno l'istituzione del Fondo nazionale per la non autosufficienza. Ancora, tra i provvedimenti di cui è stata prima firmataria, merita certamente un ricordo il disegno di legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, disegno di legge, che grazie al suo appassionato impegno, è stato approvato divenendo la legge 3 marzo 2009, n. 18, portando così a compimento l'importante lavoro svolto durante la sua esperienza di Governo nel corso della XV legislatura. Di Franca va ricordato anche l'attaccamento e l'amore per la sua città natale, per Venezia. Durante le lunghe discussioni che abbiamo avuto, ad esempio, sul tema della riforma dei porti, si è battuta con ostinazione e con grande impegno per spiegarci che Venezia aveva diritto ad una legislazione speciale, essendo il porto di Venezia, per l'appunto,

nonostante fossero ben visibili i segni della malattia, garantì sempre la sua presenza, il suo contributo lucido e propositivo ed il suo impegno ad elevare la qualità della produzione legislativa. Anche per questi motivi, signora Presidente, il suo ricordo resterà indelebile nella memoria di tutti noi, che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla e di stimarla. il 1° gennaio è morta la senatrice Cecilia Donaggio, per noi tutti Franca. Ha ceduto dopo una lunga battaglia ad un male incurabile, contro il quale ha combattuto con la tenacia e la forza proprie del suo carattere. Tutti noi la ricordiamo infatti quando, più di un anno fa, (lo raccontava anche il presidente Schifani poco fa), ritornò in Senato accolta da un grande applauso corale, dopo aver fermato in modo assolutamente imprevedibile la malattia che poi l'ha sconfitta. Della senatrice Donaggio voglio raccontare, da donna, anche alcuni tratti di storia minima, che rappresenta una base essenziale, spesso in ombra, della personalità. Franca è nata a Venezia, da famiglia operaia, socialista, quando essere socialisti non era un segno di potere, ma una difficoltà per il lavoro. Il padre operaio del vetro, la madre casalinga, due sorelle, una famiglia semplice dalla vita difficile. Franca ha raccontato tante volte la sua infanzia tra le calli veneziane dove ai bambini non si insegnava a nuotare per tenerli lontani dall'acqua. Raccontava quando un giorno, a cinque anni, la trovarono arrampicata in un campiello sulla statua di Garibaldi, in alto, senza che nessuno avesse capito come poteva esserci arrivata. Raccontava della mensa semplice, quasi povera, dove l'animale cresciuto e nutrito per Natale non veniva poi sacrificato, proprio perché in tutti era comunque presente un segno di rispetto e di civiltà. Franca è uscita con la forza di volontà dalle ristrettezze di quella realtà, ha lavorato all'ENEL, si è laureata in scienze politiche, è diventata dirigente di peso nella CGIL provinciale e regionale del Veneto, e poi nazionale. Socialista lombardiana e riformista, è stata responsabile nazionale del coordinamento donne della CGIL ed in quella qualifica l'ho incontrata per la prima volta nel 1988 a Senigallia al convegno «Quando lo Stato è donna». È stata Presidente del *Comité des Femmes* della Confederazione europea dei sindacati, è stata consigliera del CNEL, segretaria nazionale della Federazione italiana del sindacato trasporti. È stata rappresentante della CGIL nel Comitato nazionale pari opportunità presso il Ministero del lavoro e nella Commissione nazionale pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Da socialista e da riformista ha scelto poi i Democratici di Sinistra ed è stata chiamata da Piero Fassino al ruolo di vice responsabile nel Dipartimento lavoro. Ha scelto poi, con tutti noi, di entrare nel Partito Democratico, membro dell'Assemblea nazionale e della Direzione. È stata anche donna di governo, e nel maggio 2006 ha avuto l'incarico di Sottosegretario di Stato al Ministero della solidarietà sociale del Governo Prodi, con le deleghe al volontariato, all'associazionismo, alle politiche per gli anziani, all'inclusione e alla coesione sociale, alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, settore quest'ultimo che aveva sempre seguito affiancando in modo significativo, in Veneto e nel Paese, il lavoro costruito e portato avanti nel partito e nelle istituzioni dalla senatrice Anna Maria Serafini. Sul versante dei diritti dei disabili ha tra l'altro contribuito all'istituzione del Fondo per la non autosufficienza e il 30 marzo 2007 ha sottoscritto a New York la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Franca è entrata in quest'Aula come senatrice nel 2008, eletta nelle liste del Partito Democratico del Veneto e, anche in questa veste, ha continuato a mantenere un indissolubile legame con il mondo del lavoro e con il suo territorio. Oltre ai tanti disegni di legge presentati, che ripresenteremo e porteremo avanti a suo nome nella prossima legislatura, voglio ricordare qui in particolare due interventi che l'hanno vista protagonista quando già combatteva tenacemente la sua battaglia contro il cancro. Mi riferisco all'intervento pronunciato nel marzo 2012 nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro sul tema delle cosiddette morti bianche e sopratutto l'intervento, l'ultimo in Aula, del 18 luglio scorso. Franca parlava delle donne e delle loro lotte politiche. Ricordava le storiche e faticose conquiste (che mi sembra adesso si dovrebbero ricordare con un po' più di attenzione) del diritto di voto e della rappresentanza di genere. Si batteva ancora oggi per la presenza delle donne nelle istituzioni, un tema che ha segnato tutta la sua vita. Cito un piccolo brano del suo intervento: «Oggi i grandi Partiti e i grandi sindacati hanno regole che non sono più le quote di tutela, ma sono norme antidiscriminatorie: nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore o inferiore a una certa soglia. Siamo andati oltre la norma di tutela. Guardate bene le grandi organizzazioni: ci sono donne che dirigono la CGIL e la Confindustria, cose che non si sarebbero mai pensate. Ma perché, se è vero che le donne sono riuscite ad entrare in maniera così determinata nel governo anche delle grandi organizzazioni sociali, non sono mai riuscite a scalfire la politica? Gli uomini pian piano sono arretrati e oggi li vediamo asserragliati in quella che io chiamo la cittadella del potere, in cui sono loro a determinare le regole. Perché una donna non è mai stata Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e neppure Presidente del Senato? Ma la cittadella del potere non regge più. Anche quella è destinata a crollare, perché il protagonismo delle donne, non solo di quelle della mia generazione, ma anche di quelle delle giovani generazioni, spazzerà via questo atteggiamento di conservazione. Oggi, infatti, le donne vogliono sentirsi cittadine a tuttotondo. Il fatto di introdurre norme che non solo promuovano ma garantiscano anche il risultato significa solo guardare in faccia il Paese. (...) Vi chiedo solo di fare uno sforzo di modernizzazione». Cara Franca, nel chiudere anche a nome del nostro Gruppo, questo mio ricordo nell'Aula prestigiosa del Senato, voglio tenere insieme tante cose che credo i colleghi potranno comprendere: il valore del ruolo delle istituzioni che tu hai sempre saputo riconoscere e servire, il valore e il ruolo della battaglia politica in difesa dei più deboli che ha segnato tutta la tua vita dal sindacato al Partito, il valore della battaglia per i diritti delle donne, il valore dell'affetto degli amici, delle amiche, dei tuoi cari. Per la tua famiglia, che saluto, qui nelle tribune, sei stata sempre un punto di riferimento solidissimo nelle lunghe e difficili battaglie di una vita complessa. Tutte conoscevamo le storie e le vittorie professionali dei tuoi diversi nipoti, fino al più piccolo, Alvise, che abbiamo visto crescere nei tuoi racconti, fino all'iscrizione all'università che tanto ti inorgogliva. Di te resterà in noi, come ricordava Piero Fassino nel suo intervento nella Chiesa di Mira il 5 gennaio, il sorriso aperto e l'interloquire in veneto che tante volte serviva a sdrammatizzare qualche emergenza. Ancora un saluto, dunque, con l'affetto di sempre, nella certezza che le battaglie per la difesa dei diritti dei più deboli le continueremo con tenacia e le porteremo avanti anche a nome

Il pericolo è sempre quello di cadere nella retorica, ed è il motivo per il quale non me la sono mai sentita, durante tutta la legislatura, di intervenire in occasioni come queste. L'ho voluto fare oggi, personalmente, per ricordare una persona con cui ho lavorato nella Commissione lavori pubblici. Non voglio quindi ripercorrere la sua biografia: l'ho letta, ieri mi sono documentato su quello cha ha fatto nella sua vita personale, professionale e politica Franca Donaggio, ma ritengo che andrei a ripetere quanto hanno già detto persone prima di me sicuramente molto meglio di quanto sarei in grado di fare io oggi. Voglio, però, ricordare la collega; una collega con le idee molto distanti dalle mie. Infatti, era consuetudine anche beccarsi un poco. Avevamo posizioni sicuramente molto, molto distanti dal punto di vista politico e ideologico, ma era veramente veramente bello confrontarsi sui temi importanti della vita di tutti i giorni, della vita della nostra gente, partendo da due visioni completamente opposte, per poi arrivare a scoprire che la base da cui partiva la passione del fare politica e dell'impegno era assolutamente la stessa: amore per la propria terra, amore per la propria gente, amore per i valori

che metterò nel mio bagaglio di esperienze personali e anche politiche di questa legislatura

un po' ironico, che utilizzava per il confronto con me, per esempio, che ero distantissimo dalle sue posizioni: lo stesso sorriso ironico che ha utilizzato per

Presidente, dopo gli interventi dei colleghi, intendo esprimere una riflessione sulla collega Donaggio, con brevità, ma con intensità e con partecipazione emotiva. Chissà perché, pensando alla senatrice Donaggio, mi viene in mente una canzone di Ligabue: «Una vita da mediano», in quanto esprime e simboleggia la tenacia, la determinazione, la solidità, la capacità di fare squadra, doti e valori che fanno il profilo e lo stile di una persona. A me pare che il profilo e lo stile della collega Donaggio fossero improntati a questi valori: alla tenacia, alla determinazione, alla solidità, alla capacità di fare squadra. squadra. Abbiamo bisogno di ricordare figure che appartengono a quel lavorio oscuro, a volte impersonale, che però è così significativo, così importante, perché dà senso e dignità alla politica, perché dà senso ed umanità alla politica. Ho conosciuto la collega Donaggio non solo nell'esperienza parlamentare: l'ho conosciuta da Sottosegretario (prima lo sono stato io, poi lei, poi ancora io), quando abbiamo avuto rapporti di collaborazione improntati alla cooperazione istituzionale al di là delle appartenenze, ed ho sempre trovato una persona aperta al confronto e al dialogo, pur nella consapevolezza dei suoi principi, dei suoi valori, dei suoi convincimenti. Ecco perché la ricordo con nostalgia; ecco perché dico che la collega Donaggio è stata davvero una bella persona e davvero una bella collega. esprimiamo alla sua famiglia ed al Gruppo del Partito Democratico piena solidarietà nel suo ricordo, nel suo insegnamento, che credo abbia trovato oggi nell'Aula del Senato il giusto riconoscimento.

Signora Presidente, andando a leggere la nota biografica relativa a Cecilia Donaggio (a Franca Donaggio)

Mi sembra un atto di orgogliosa rivendicazione, che noi siamo in grado di apprezzare, che la colloca su un piano volutamente espressivo: sono dirigente politico, ma per ciò stesso sono fuori dalla casta. La senatrice Donaggio era fuori dalla casta: era una dirigente politica che era cresciuta nelle lotte del movimento operaio e che si è sempre battuta sul terreno dei diritti del lavoro, dei diritti umani, dei diritti dei più deboli. Ed è arrivata in Parlamento giustamente, perché in Parlamento dovrebbero arrivare persone così, forse di più di quelle che ci arrivano normalmente. Era un esempio di serietà, di sobrietà, senso della misura e capacità anche di incidere, in senso disciplinare, sui temi che trattava. Penso che la senatrice Donaggio fosse un esempio di ottimo parlamentare, senza troppe chiacchiere, senza sbavature e con la capacità di riuscire a produrre un effetto conforme allo scopo, all'azione che svolgeva.

È scomparsa per lungo tempo, abbattuta dalla malattia, e quando è ritornata era asciugata, assottigliata dalle cure e dalla stanchezza della malattia; all'inizio - lo confesso - per certi aspetti era perfino irriconoscibile, però gli occhi e il sorriso erano gli stessi di prima e parlavano come prima. La senatrice Donaggio è un esempio di parlamentare che ricordiamo con affetto, l'esempio di come si deve essere dentro quest'Aula. Le tributiamo pertanto un saluto affettuoso e la porteremo a lungo nella nostra memoria.

ha lottato contro una terribile malattia, eppure, nonostante le pesanti terapie alle quali era costretta, fino all'ultimo ci ha onorato della sua presenza in quest'Aula, con la dedizione ed il senso del Governo che le appartenevano. Nonostante la malattia, non ha mai perso l'attenzione per il suo ruolo e la sua città, e il suo impegno ed il suo contributo non sono mai venuti meno. Ritengo una fortuna e un privilegio averla conosciuta, averle sorriso ed aver ricevuto il suo sorriso, fino all'ultimo. La militanza in opposti schieramenti non ha mai fatto venir meno il rispetto reciproco e, da parte mia, l'ammirazione e l'apprezzamento per la sua capacità di lavoro, la sua tenacia e la determinazione con le quali ha portato avanti le sue battaglie, spesso condivise, sui temi del lavoro e dell'uguaglianza sociale. Con lei scompare un'altra donna, un'altra figura di donna forte e coraggiosa. Nel mondo del lavoro prima, con l'esperienza nella CGIL, e nella politica poi, Franca Donaggio ha lavorato alla ricerca di politiche inclusive a sostegno delle categorie più disagiate. Una donna forte, sempre pronta a dar voce alle richieste e alle esigenze dei più deboli, costantemente in prima linea nelle battaglie a favore delle donne, dei lavoratori e dei precari. Ricordo anche il suo contributo come Sottosegretario alla solidarietà sociale nel secondo Governo Prodi, nel 2006, e nell'istituzione del Fondo per la non autosufficienza. Franca è stata un esempio per tutti noi: un esempio di vita e d'impegno politico, lo dico con il cuore, non in maniera formale. Noi del Gruppo Fratelli d'Italia, ma penso anche tutti gli altri, non la dimenticheremo: ciao, Franca!

ritornano alla mente i momenti significativi, in cui le reciproche vite si sono incontrate e incrociate. Per questo motivo, nel rammentare Franca Donaggio la solidità morale e l'onestà intellettuale, la passione e l'esperienza

l'esperienza vissuta insieme a lei come componente della Commissione per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi donne abbiamo avuto una grande fortuna, perché abbiamo vissuto questo grande momento d'incontro e confronto proprio in quella Commissione. Per me si trattava dei primi passi in politica, pertanto quello è stato un passaggio fondamentale all'inizio della mia vita politica: da Franca Donaggio ho imparato molto, perché con lei sono riuscita a costruire un rapporto forte, leale e creativo, che ci ha spinte a cercare e creare sempre un punto d'incontro su ciò che ci univa. L'esperienza di quella Commissione ha segnato il percorso di molte di noi e ha costituito, soprattutto, la base di tanti dibattiti che sarebbero poi stati ancora al centro nel Paese e nelle Aule parlamentari, sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni,

che ci portiamo dietro dall'inizio del Novecento». In quell'appassionato intervento terminava dicendo: «Vi chiedo solo di fare uno sforzo di modernizzazione. Guardate in faccia le nuove generazioni delle donne.

in cui le donne fecero una battaglia per la rappresentanza femminile nelle più alte cariche istituzionali». Ecco, finisco con questa affermazione, perché credo che queste parole di grande densità politica e qualità civile debbano essere l'obiettivo comune di tutti, uomini e donne. Signora Presidente, la ringrazio per avermi voluto concedere la possibilità di lasciare traccia di un mio pensiero dedicato a Franca Donaggio. Aggiungo alle parole importanti che sono risuonate in questa Aula le mie modeste parole: parole di chi ha conosciuto Franca, l'ha conosciuta lungo una vita che, come il senatore Pardi ha detto benissimo prima, è stata, sempre, in tutti i suoi giorni, il compimento di un atto politico. La sua vita e la sua morte sono, infatti, per me un atto politico, per il segno indelebile che lascia Franca nella storia delle donne italiane e per la gratitudine che le donne italiane debbono ad una donna come Franca Donaggio, che ha sempre anteposto al suo interesse personale e alla sua vita stessa, la vita, la storia e la difesa delle donne e di chiunque fosse in una condizione di difficoltà e di disagio, per realizzare quel principio di pari opportunità garantito dalla nostra Costituzione, ma che non sempre riusciamo a tradurre in atti concreti. La vita e la concretezza di Franca Donaggio sono per noi una testimonianza e, per tante di noi, per chi ha avuto la fortuna di conoscerla e anche per chi magari non l'ha avuta, un modello di donna da seguire.

recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione***

onorevoli colleghi, il decreto al nostro esame reca, giustamente, la proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace e ai connessi interventi di cooperazione civile. La proroga copre il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013 (nove mesi, anziché un anno come nel 2012). Le ragioni di questo cambiamento sono da imputare all'entità delle risorse finanziarie predisposte dal Governo per il 2013. Lo stanziamento complessivo ammonta a 935 milioni di euro. Viene quindi utilizzato quasi interamente il rifinanziamento del fondo missioni (1.004 milioni di euro) disposto dal decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012. Una somma significativamente inferiore a quella stanziata l'anno precedente (1.403 milioni) per un periodo di 12 mesi. Il decreto-legge in esame è l'ultimo atto di questo genere che viene adottato nella XVI legislatura. È l'atto normativo che probabilmente segna anche la fine dei lavori del Senato alla vigilia della campagna elettorale. Gli anni della corrente legislatura sono stati pieni di sfide e di significative evoluzioni degli scenari d'impegno delle Forze armate italiane nelle aree più delicate del pianeta. Sottolineo come su questi impegni si sia sempre registrata un'ampia convergenza delle forze politiche di maggioranza e dì opposizione. Un segno questo che conferma il pieno sostegno del Parlamento all'azione dei nostri militari e civili, nel solco dei principi chiaramente fissati nella Costituzione repubblicana. Lasciando all'esposizione del relatore per la Commissione difesa, senatore Del Vecchio, il compito di illustrare gli impieghi nelle singole missioni, mi limito a richiamare la missione più significativa, quella in Afghanistan, che assorbe 426 milioni di euro, cioè quasi la metà dello stanziamento complessivo. Ci si avvicina al 2014, anno in cui è fissata la transizione per il passaggio dei poteri alle autorità afghane e il disimpegno militare della missione ISAF. Da quel momento in poi la presenza della NATO sarà focalizzata sulle attività di formazione e assistenza alle forze di sicurezza nazionali, titolari delle responsabilità sulla situazione del Paese, garantendo da parte nostra un sostegno finanziario previsto in misura significativa fino al 2017. La transizione dovrà presumibilmente essere accompagnata da un processo di riconciliazione nazionale che richiede, oltre alla stabilizzazione dell'area, anche un dialogo politico con l'insorgenza. Sarà un processo a guida locale che auspicabilmente dovrà portare alla rinuncia alla violenza, a combattere più efficacemente la corruzione, alla rottura dei legami con il terrorismo internazionale, riconoscendo princìpi fondamentali quali la tutela dei diritti umani e il rispetto della parità di genere, delle donne e dei bambini. Mi soffermerò ora sul Capo II del decreto-legge, che è di specifica competenza della Commissione affari esteri. Esso prevede la partecipazione a iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno alla ricostruzione per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. Lo stanziamento complessivo per tali attività è di 81 milioni di euro, meno del 10 per cento del totale di spesa autorizzato. L'articolo 5 del provvedimento autorizza la partecipazione a iniziative e interventi di cooperazione allo sviluppo in Afghanistan (15 milioni di euro), Pakistan, Iraq, Libano, Libia, Myanmar, Somalia, Sudan e Sud Sudan (20 milioni di euro), integrando gli stanziamenti già assegnati dalla legge di stabilità del 2012 e dalla legge n. 49 del 1987, oltre che dai programmi di sminamento umanitario per i quali è previsto uno stanziamento di 500.000 euro. Lo scenario più impegnativo è nuovamente quello dell'Afghanistan, dove lo stanziamento che ho ricordato di 15 milioni di euro è assicurato dal rifinanziamento della legge n. 49 del 1987, che è rivolto anche ad iniziative indirizzate al Pakistan. L'Italia è chiamata ad adempiere gli impegni assunti come stabiliti nella Conferenza di Tokyo del 9 luglio 2012, riguardanti in gran parte le prospettive di ricostruzione dell'Afghanistan successivamente al ritiro di ISAF. L'erogazione degli stanziamenti avverrà attraverso il canale bilaterale e multilaterale, con interventi umanitari e di emergenza e per il tramite delle ONG. Per quanto concerne i rapporti bilaterali, ricordo che il 26 gennaio 2012 il presidente Karzai, in visita a Roma, ha firmato a nome della Repubblica islamica dell'Afghanistan un accordo con la Repubblica italiana sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra i due Paesi, accordo ratificato dal Senato il 30 ottobre 2012. Ricordo che il presidente del Consiglio Monti si è recato in visita in Afghanistan il 4 novembre dello scorso anno e in tale occasione ha ribadito il sostegno italiano anche dopo il 2014, spostando l'attenzione dal versante militare a quello economico e della *capacity-building*. Di interesse è la cooperazione economica prevista per il Myanmar, Paese che sta affrontando un processo di apertura e di sviluppo socio-economico inclusivo. Particolare attenzione verrebbe inoltre dedicata alla Siria e ai Paesi limitrofi, sostenendo le istituzioni internazionali che tutelano il patrimonio culturale e la salute dei cittadini e assistono, anche dal punto di vista sanitario, i campi profughi particolarmente esposti a violenza e insicurezza. L'articolo 6 del decreto riguarda il sostegno ai processi di ricostruzione e stabilizzazione nelle aree di grave conflitto e instabilità sociale quali Afghanistan, Iraq, Libia, Siria e Yemen. Al riguardo il decreto prevede il finanziamento dell'Italia ad iniziative delle organizzazioni internazionali, compresa la partecipazione ai fondi fiduciari della NATO (per 1,45 e ai programmi dell'Unione europea nel campo della gestione delle crisi in ambito PESC-PSDC (per 3,039 nonché dell'OSCE (570.000). Sono previsti interventi operativi in questi Paesi per la tutela dei cittadini italiani e degli interessi italiani (per uno stanziamento di oltre 16 milioni), per per il rafforzamento delle strutture delle sedi diplomatiche nei territori ad elevato rischio (per 4,5 milioni) e per la loro messa in sicurezza (per 9,5 milioni). Stamani, nell'audizione con gli onorevoli Ministri degli esteri e della difesa, il ministro Terzi di Santagata ha sottolineato quanto sia importante rendere sicure le nostre sedi diplomatiche in aree di crisi. Quanto alla Libia, le operazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 6 prevedono la prosecuzione della formazione per il controllo dei flussi di merci e di persone attraverso la frontiera libica, con un finanziamento di euro 800.000 e la formazione nel settore dei media, e quindi dei giornalisti, (per 200.000), oltre al ripristino della funzionalità dell'Istituto italiano di cultura a Tripoli (78.000). Ricordo che nella giornata di giovedì 10 gennaio le Commissioni esteri del Senato e della Camera hanno incontrato il Presidente del Congresso Nazionale e Capo provvisorio dello Stato della Libia, Mohammed Magariaf (accompagnato da un'ampia delegazione governativa), il quale ha riaffermato che l'Italia e la Libia sono legate da vincoli storici e culturali indissolubili.

che minano la stabilità stessa del Paese. Le autorità sono ora impegnate in un profondo processo di riforma democratica delle istituzioni. costituisce la premessa indispensabile per lo sviluppo economico e per il pieno inserimento della Libia nello scenario europeo, mediterraneo ed internazionale. Con profondo rammarico sottolineo che, dopo le preoccupazioni espresse dal presidente Magariaf durante la sua visita a Roma circa l'insicurezza che regna ancora nel Paese, nella serata di sabato 12 gennaio è avvenuto il vile e brutale attentato al console d'Italia a Bengasi, fortunatamente rimasto illeso insieme alla sua scorta, grazie alla blindatura del loro mezzo, e a seguito del quale il Governo, esprimendo la più ferma condanna, ha disposto la chiusura temporanea del consolato stesso. Rispetto alla Siria, il decreto prevede un sostegno ai processi di ricostruzione e di stabilizzazione che dovrebbe essere meglio finalizzato nel decreto per evitare ambiguità. L'articolo 7 prevede poi disposizioni che disciplinano il regime degli interventi civili, con una novità (al comma 11) che consente ai coniugi del personale militare e civile destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero di fruire di un limitato periodo di collocamento in aspettativa, sia nell'ambito pubblico che privato, come avviene per i coniugi dei funzionari di organizzazioni internazionali.

all'intervento in Siria. Gli stessi senatori avevano presentato al riguardo il disegno di legge n. 3458, il cui disposto dunque si potrebbe considerare sostanzialmente assorbito dal provvedimento in esame. Insieme al relatore Del Vecchio ho predisposto emendamenti che apportano mere modifiche di *drafting* al testo del decreto-legge. si propone l'approvazione da parte del Senato del disegno di legge che si inquadra nell'ambito della partecipazione dell'Italia ad importanti operazioni di mantenimento della pace e della sicurezza e nella stabilizzazione di aree di crisi in contesti geografici molto difficili. Signora Presidente, come Presidente della 3a Commissione permanente - credo che farà altrettanto il senatore Del Vecchio - ho tenuto a fare una presentazione dettagliata del provvedimento in esame perché è di difficile lettura, essendo costituito da 300 pagine (sono certo che non tutti i senatori lo hanno potuto esaminare).

le missioni internazionali di cui oggi esaminiamo la proroga sono state oggetto di un confronto nello scorso mese di ottobre tra il Governo e le Commissioni esteri e difesa della Camera e del Senato. Il decreto alla nostra attenzione traduce quindi in oneri di spesa le conclusioni del dibattito avvenuto in quella circostanza. Le missioni da rifinanziare sono esplicitate nell'articolo 1 del decreto e possono essere suddivise in due blocchi. Tra le operazioni di maggiore impegno va innanzitutto menzionata quella in Afghanistan, che comprende la missione ISAF della NATO, per il sostegno del Governo afghano nel controllo del territorio, e la missione EUPOL dell'Unione europea, finalizzata alla formazione delle forze di sicurezza locali. All'impegno nel Paese asiatico è associato, per i primi nove mesi del 2013, un onere di spesa pari a circa 426 milioni di euro, sensibilmente inferiore (di circa 150 milioni) a quello sostenuto per lo stesso periodo nel 2012, grazie alla riduzione del personale militare impiegato, dalle 4.000 unità in conseguenza del progressivo passaggio del controllo dei distretti del Paese dalle forze internazionali a quelle locali. Nel settore di interesse dell'Italia questo passaggio è già avvenuto a Bala Murghab, nel Gulistan, ed a Bakua ed avverrà nel corrente anno ancora a Bala Baluk e Farah. Altra missione di rilievo è l'operazione UNIFIL in Libano, che comporterà per i primi nove mesi dell'anno in corso una spesa di circa 119 milioni di euro.

In merito a questa missione, che è la più importante tra quelle gestite direttamente dall'ONU, giova ricordare che la *leadership* è ancora una volta italiana e che la carica di comandante di tutte le forze internazionali è ricoperta dal generale Serra. Vanno quindi considerate le operazioni nei Balcani, rappresentate dalla *Multinational* *specialized* *unit* (MSU), dalla missione Eulex e dall'operazione *Joint enterprise*. In questo caso, in relazione al progressi del processo di stabilizzazione dell'area, è stato possibile ridurre il personale impiegato da 850 a 470 unità, contenendo sensibilmente gli oneri finanziari. un cenno alle operazioni navali nel Mediterraneo e al largo della Somalia, che comprendono le missioni *Active Endeavour* e *Ocean Shield* della NATO e la missione Atalanta dell'Unione europea. Le finalità di queste operazioni sono la prevenzione e la protezione contro azioni terroristiche e di pirateria marittima. Gli oneri finanziari relativi ammontano a circa 48 milioni Anche in questo caso va sottolineato il fatto che il comando dell'operazione *Ocean Shield* è attribuito all'Italia, con l'ammiraglio Natale. Oltre alle operazioni di maggior rilievo che ho finora ricordato, sono previste altre 17 missioni ed attività. Nella quasi totalità dei casi, queste operazioni di minor impatto finanziario sono state avviate negli anni passati e non presentano sostanziali modifiche. Tra di esse, peraltro, merita di essere menzionata l'operazione dell'Unione europea denominata Sahel Niger. Quest'ultima operazione è diretta a sostenere le autorità nigeriane nello sviluppo di una strategia di sicurezza nell'area centrale dell'Africa, con riguardo anche ad iniziative per la formazione delle forze di sicurezza del Mali. In merito alla situazione nel Mali, il recente intervento aereo francese contro gruppi di criminali e terroristi nel Nord del Paese ha determinato una improvvisa evoluzione che sarà oggetto d'esame in un vertice dei Ministri degli affari esteri dell'Unione europea convocato per domani. Sono pertanto possibili nuove iniziative della comunità internazionale e coinvolgimenti dei Paesi europei per la sicurezza dell'area, tenuto anche conto della risoluzione dell'ONU n. 2085 del 20 dicembre 2012 che autorizza l'avvio di una missione a *leadership* africana per la stabilizzazione del Paese, missione che peraltro non è ancora iniziata. L'articolo 1, di cui ho finora riferito, reca altre importanti autorizzazioni di spesa. Vorrei in questa sede ricordare quella concernente gli interventi dei contingenti militari per assicurare le prime necessità alle popolazioni in Afghanistan, in Libano, nei Balcani e nel Corno d'Africa, per i quali sono state previste risorse per 6,5 milioni di euro. Riepilogando quanto previsto all'articolo 1, gli oneri finanziari complessivi delle missioni, per il periodo di nove mesi, sono pari a circa 853 milioni di euro, a cui vanno aggiunte le risorse di cui ha già parlato il senatore Dini per un totale di 935 milioni di euro. Nell'articolo 2 trovano collocazione disposizioni in materia di indennità da erogare al personale impiegato nelle missioni e di trattamento assicurativo e pensionistico. Queste disposizioni sono analoghe a quelle applicate negli anni passati. stesso articolo sono presenti norme che, traendo spunto dalle esigenze delle missioni, consentono alla Polizia di Stato sia di assumere agenti di polizia, sia di attivare procedure concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovraintendente; in sostanza, norme che avviano il superamento del blocco del *turnover.* Nell'articolo 3 sono ribadite le disposizioni in materia di disciplina penale militare per coloro che operano nelle missioni internazionali. In particolare sono confermati il codice penale militare di pace, la competenza territoriale del tribunale militare di Roma e la scriminante in tema di uso legittimo della forza, quale tutela sul piano giuridico per il personale militare. militare. L'articolo 4 reca infine disposizioni in materia contabile. La più importante di queste disposizioni è quella che prevede la rapida anticipazione

L'entità complessiva del personale militare e di polizia impiegato si attesta sulle 6.000 unità. È un livello inferiore a quello di alcuni anni fa, quando furono raggiunte e superate le 12.000 unità, ma ciò è conseguenza delle note difficoltà finanziarie del Paese che impongono valutazioni oculate sul livello di partecipazione alle operazioni di stabilizzazione. Comunque, pur nel quadro della suddetta contrazione delle forze, l'Italia continua a esercitare un ruolo significativo nei processi di pace e di superamento delle crisi internazionali. Infatti è presente nelle missioni di stabilizzazione che si svolgono in 14 Paesi diversi; opera, con i propri contingenti, nei teatri operativi più delicati (Vicino e Medio Oriente, Africa settentrionale e centrale, penisola balcanica ed Europa orientale, Mar Mediterraneo e Oceano Indiano); detiene, come prima sottolineato, la *leadership* della missione ONU in Libano, che è determinante per evitare l'aggravamento delle crisi nell'area, e di quella navale «*Ocean Shield*», per il contrasto della pirateria; fornisce un contributo di forze complessivo, confrontabile con quello dei principali Paesi europei per le operazioni NATO ed Unione europea e superiore a quello degli stessi Paesi per le operazioni sotto l'egida dell'ONU; esprime infine una peculiare capacità di svolgere le delicate funzioni di stabilizzazione, che è unanimemente apprezzata. L'ultima notazione è relativa ad un principio che costituisce da sempre la base della partecipazione del Paese alle operazioni internazionali. L'impegno dell'Italia continuerà nel 2013 esclusivamente in missioni che coinvolgono gli interessi nazionali nel settore della sicurezza ma che mantengono la più alta legittimazione internazionale, in quanto promosse o condotte su mandato dell'ONU, dell'Unione europea o della NATO. Per le ragioni che ho appena evidenziato e ringraziando tutti i connazionali, militari e civili, che operano per la pace e la stabilizzazione delle aree di crisi, spesso a rischio della propria incolumità, anch'io propongo come il presidente Dini, l'approvazione da parte del Senato del provvedimento relativo alla proroga delle missioni internazionali.

Ci sono però alcuni argomenti sui quali credo sia opportuno concentrare almeno da parte nostra l'attenzione. Alcuni possono essere argomenti di carattere formale, ma

andavano verificate con una certa frequenza, proprio per dimensionare al meglio gli interventi e le azioni delle nostre Forze armate all'estero. Aver prorogato le credo denunci un modo non corretto di gestione della cosa pubblica. È evidente che il Governo si è trovato di fronte alla necessità di coprire una spesa che nella legge di stabilità non aveva copertura.

ci sforziamo di cercare un consenso all'interno del Parlamento che sia superiore alle parti di maggioranza e minoranza proprio per dare maggiore forza e credibilità all'azione dei nostri militari, credo che l'aver usato questo metodo dei nove dodicesimi

l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge, che prevede un'autorizzazione di spesa di 3.948.000 euro per interventi a sostegno di processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, conflitto o *post* conflitto.

per un'esigenza di natura contabile (sappiamo ormai quanto conti la Ragioneria dello Stato e la logica ragionieristica anche nella scrittura delle leggi),

a quelle che saranno le operazioni dell'auspicato *day after* dopo la caduta di Assad. Ora, francamente questo mi sembra un *unicum* nelle relazioni internazionali. internazionali. Capisco le esigenze contabili, ma credo ci siano anche le esigenze della politica e dei buoni rapporti internazionali. Non chiedo molto: con l'ordine del giorno G6.100, che invito i colleghi a sottoscrivere e votare, desidero impegnare il Governo ad individuare finalizzazioni per gli interventi italiani di ricostruzione riferiti ad interventi straordinari in Siria più conformi alla situazione in atto e ai suoi possibili sviluppi, modificando ovvero integrando i documenti tecnici di accompagnamento al decreto‑legge. Vorrei inoltre sapere dal Governo se il Parlamento siriano indicato nella relazione tecnica è è quello attuale, cioè l'unico legittimo Parlamento siriano (si può discutere nel merito, ma tale è per la legge internazionale), oppure se già prevediamo gli aiuti al prossimo Parlamento.

Colgo l'occasione per dire al Governo che forse, in sede europea, occorrerà anche prendere una posizione molto precisa. Ora, non voglio Ora, non voglio qui fare polemica sull'intervento francese e sugli articoli di Bernard-Henri Lévy che sembra essere diventato il messaggero di pace della Francia repubblicana e imperiale. Lasciamo perdere la polemica con gli alleati francesi e con i nostri *partner* d'Europa.

Ci sono ragioni sociali, storiche ed etniche. Quando si parla dei Tuareg vorrei ricordare che sono berberi e non arabi e in quell'area l'appartenenza all'una o all'altra delle due etnie non è priva di significato, anche se sono poi unite nella religione islamica. Così come il problema specifico del Mali non è nemmeno un problema nuovo. Voglio ricordare che i Tuareg si sono sollevati ben tre volte contro il Governo centrale maliano in questo momento l'area occupata dai ribelli corrisponde alle rivendicazioni nazionaliste dei Tuareg. Occupano infatti un territorio del Mali, tanto per dare un'idea, che è grande come la Francia

Siamo quindi in una situazione che non è di contrasto politico o di orientamento ma è radicata nella storia, nel tempo e nei costumi e quindi va politicamente affrontata. L'azione militare non può che essere una risposta all'emergenza temporanea per evitare che, al di là dei confini di quella che i Tuareg ritengono sia l'area di loro competenza, crolli sostanzialmente il regime maliano e vi siano ovviamente situazioni particolari, qualora le colonne armate della rivoluzione Tuareg dovessero arrivare a Bamako. L'invito che rivolgo al Governo italiano che siederà al tavolo con i *partner* europei è quindi quello di non cadere nella trappola delle emergenze, che poi finisce lì con l'intervento militare. Occorre aprire un grande dialogo e dibattito all'interno dell'Unione europea

Occorre cioè auspicabilmente avviare un grande processo politico di dialogo, utilizzando anche l'incaricato speciale delle Nazioni Unite, che è il professor Prodi, che peraltro si sta impegnando molto su questa vicenda. Occorre quindi riprendere questa iniziativa e far allontanare da tutti noi l'idea che l'intervento francese sia un intervento nella ex colonia del Mali con una predominanza di una parte dell'Europa (è già avvenuto qualcosa di analogo in Costa d'Avorio, e chiudiamo la partita, per carità d'Europa).

generale dello Stato in materia di copertura e di definizione dei fondi, ma che riprenda un'iniziativa politica nel Nord dell'Africa che abbiamo interrotto da qualche tempo in qua.

Presidente, colleghi, come avviene in occasione di ogni conversione dei decreti-legge recante la proroga delle missioni internazionali, l'Italia dei Valori non può che esprimere alcune perplessità concernenti, principalmente, la questione relativa all'Afghanistan e l'impegno che il nostro Paese ha assunto in quell'area del Prima di arrivare, però, a disquisire di quanto appena citato, vorrei fare una breve panoramica del decreto evidenziando i punti che riteniamo essere condivisibili e quelli che, invece, a nostro giudizio, meritano qualche ulteriore riflessione. Abbiamo innanzitutto notato come il presente decreto, a differenza del precedente, non disponga la proroga annuale delle missioni, ma abbia, bensì una copertura fino al 30 settembre 2013. Per evidenti motivi, legati innanzitutto alla natura di questo Governo e alla fine della legislatura, comprendiamo e condividiamo tale scelta. Non possiamo, però, esimerci dall'auspicare che la prossima legislatura dia vita ad una legge quadro che disciplini le missioni internazionali e il nostro impegno fuori dai confini nazionali. Questa precarietà non rende giustizia, né a chi lavora nei teatri operativi esteri, né ai Paesi con i quali e nei quali interveniamo. Come poi rilevato anche da autorevoli colleghi durante l'esame svolto in Commissione, nel decreto-legge si rinvengono disposizioni che non attengono strettamente al profilo dell'impegno militare all'estero e della ricostruzione civile. Di conseguenza, è evidente la spiccata eterogeneità dei contenuti, profilo peraltro di incostituzionalità. Inoltre, ed approfitto per chiedere ragguagli al Governo in tal senso, le disposizioni e gli stanziamenti relativi sia alla Siria che al Libano appaiono non esser calibrati sulla situazione esistente. Nel dettaglio, sembrerebbe che il Governo ritenga già chiusa la partita siriana con una capitolazione del regime di Bashar al-Assad (cosa che appare tutt'altro che certa) mentre non ravvisa alcun rischio, o comunque necessità di rinforzo, di quella che da sempre è la missione più importante che l'Italia porta avanti; mi riferisco al fiore all'occhiello delle nostre missioni internazionali, sia storicamente che al momento attuale, il Libano. Questa missione, nonostante la delicatissima situazione regionale, sconta ancora, e come meglio dirò in seguito, il ricatto della Lega Nord sul precedente Governo con la decurtazione della partecipazione sia in termini finanziari, che numerici. Venendo al contenuto del decreto nel dettaglio, l'articolo 1 disciplina il nostro impegno in Afghanistan e prevede lo stanziamento di 426 milioni di euro. Rispetto a quanto stanziato nei precedenti decreti, si registra, dunque, una significativa contrazione. È sicuramente una buona notizia, ma a nostro avviso, non è sufficiente. I quotidiani, nei giorni scorsi, ci informavano che gli Stati Uniti, per bocca del vice consigliere la sicurezza nazionale Rhodes, per la prima volta, hanno paventato "l'Opzione zero", ovvero l'ipotesi di un ritiro totale delle forze militari statunitensi dopo il 2014. Persino gli Stati Uniti hanno dunque intenzione di porre fine al proprio impegno in una guerra che non ha avuto mai, né vincitori, né vinti. Noi siamo a favore, dunque, di un ritiro immediato. L'altra missione disciplinata all'interno dell'articolo 1 - come già anticipato - è quella in Libano dove si prevede una spesa di 118.540.833 euro, cifra, quest'ultima, pressoché identica a quella dell'anno precedente. A tal proposito ci saremmo aspettati, a fronte di una situazione in netto peggioramento, uno stanziamento maggiore. Le stesse Nazioni Unite hanno infatti affermato recentemente che le milizie in Libano hanno a disposizione sempre più armi e che il numero degli scontri è aumentato notevolmente (la situazione è, dunque, molto pericolosa) e invitano quindi le parti in causa a fare di più per ridurre le tensioni. Nulla in contrario, invece, relativamente alle missioni nei Balcani, nel Mediterraneo, in Somalia e a quelle di contrasto alla pirateria che avevano già, nel precedente decreto, registrato un significativo rafforzamento sia in termini finanziari, che di uomini. In generale, l'Italia dei Valori si rallegra del fatto che l'Europa abbia preso consapevolezza della situazione africana e dei rischi legati al terrorismo in questo continente. Saremo attenti a questo processo internazionale di prevenzione che speriamo non sfoci mai, come purtroppo in passato è successo, in esportazioni violente della democrazia. Per questo, sia per quanto riguarda il Niger che per il Corno d'Africa, come per la situazione in Mali, auspichiamo un confronto leale e trasparente con il Governo, perché non vorremmo ritrovarci tra pochi giorni con i nostri ragazzi ostaggi in quelle aree. Strettamente attinente all'ambito di interesse della Commissione difesa, sono gli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento che recano disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali, di norme in materia penale, nonché di norme di contabilità e modifiche al codice dell'ordinamento militare. Le novità rispetto ai decreti precedenti sono contenute nei commi 3 e 5 dell'articolo 2 e riguardano una più specifica disciplina dell'attribuzione delle indennità di missione e una deroga ai limiti delle assunzioni relativi al Corpo della Polizia di Stato. Per quanto concerne le disposizioni in materia penale, il decreto propone, invece, un rinvio normativo che prevede l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali del codice penale militare di pace e altre disposizioni verso le quali siamo abbastanza favorevoli. Nulla in contrario, nemmeno, a quanto previsto nell'articolo 4, ossia l'applicazione di disposizioni in materia contabile anche alle missioni internazionali e la possibilità Riteniamo che questa misura, fin quando non ci sarà una legge quadro che stabilizzi il nostro impegno, possa considerarsi una soluzione necessaria a garantire una certa stabilità e continuità. L'Italia dei Valori è da sempre stata favorevole all'impegno del nostro Paese nelle missioni internazionali di cooperazione. È per questo motivo che siamo favorevoli a quanto contenuto nell'articolo 5. Anche in Afghanistan, ad esempio, riteniamo che sia questo il tipo di intervento necessario e da prediligere. Una stabilizzazione dell'Afghanistan, infatti, a nostro giudizio non può avvenire per mano di una forza armata. Deve esserci un'azione internazionale volta a favorire la cooperazione e lo sviluppo del Paese. Il mio partito è favorevole al mantenimento degli impegni assunti in occasione della Conferenza di Tokyo dello Analogo discorso vale per quanto disposto nell'articolo 6, ovvero per la partecipazione del nostro Paese alle missioni di ricostruzione e consolidamento dei processi di pace. La previsione poi di costituire strutture operative temporanee nei casi di necessità e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, così come previsto all'articolo 7, risulta condivisibile. Concludo sostenendo comunque

disposto nella nostra Carta costituzionale, occorra pensare e predisporre un ritiro totale ed immediato delle Forze armate. Vorrei infine invece denunciare il depauperamento dei fondi destinati alla cooperazione.

Signora Presidente, signori Sottosegretari, onorevoli colleghe e colleghi, la proroga delle missioni internazionali oggi all'esame di quest'Aula prevede l'autorizzazione di spesa per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2013. Si parla quindi di nove mesi al posto di un anno. Lo stanziamento complessivo ammonta a 935,5 milioni di euro, con il contestuale utilizzo nella quasi totalità del rifinanziamento del fondo missioni disposto dal decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, pari a 1.004 milioni di euro. Si tratta di impegno vasto ed articolato e per quanto concerne gli aspetti di interesse della Difesa voglio evidenziare le missioni più significative che vedono impegnato il nostro Paese. In Afghanistan ci troviamo in una fase cruciale, in quanto nel 2014 è previsto il passaggio dei poteri alle autorità afghane, come confermato dal Vertice NATO di Chicago del 2012. Tale transizione dovrà essere accompagnata anche da un processo di riconciliazione nazionale, che porti alla rinuncia alla violenza e all'isolamento del terrorismo stesso. In ogni caso, il graduale passaggio di responsabilità alle autorità di sicurezza locali è percepibile anche avendo riguardo all'onere di spesa, pari a circa 426 milioni di euro, ed inferiore a quello previsto per lo stesso periodo nel 2012, a causa della riduzione del personale militare impiegato (che scende dalle 4.000 unità del 2012 alle 3.100 attuali). Il Paese si vede inoltre impegnato in una serie di altre importanti missioni internazionali: l'operazione UNIFIL in Libano, che comporterà, per i primi nove mesi dell'anno in corso, la spesa di 119 milioni di euro, e che rimane una missione fondamentale anche in relazione ai riflessi della crisi siriana; la missione nei Balcani; la Eulex in Kosovo; Joint Enterprise, ancora in Kosovo; l'operazione Althea in Bosnia, dove il personale impiegato passa da 850 a 470 unità, contenendo sensibilmente gli oneri finanziari. Non si devono poi dimenticare le importanti operazioni marittime nel Mediterraneo ed al largo della Somalia, e la missione Atalanta dell'Unione europea, che hanno la finalità di prevenire e proteggere dalle azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo ed al largo della Somalia e del Corno d'Africa. I relativi oneri finanziari ammontano a circa 48 milioni di euro, con una leggera diminuzione rispetto al 2012. Inoltre il decreto in esame prevede al suo interno altre 17 missioni ed attività, nonché altre importanti disposizioni, tra cui voglio sottolineare quelle relative alla cessione a titolo gratuito di mezzi, materiali e vestiario non più utilizzati dalle Forze armate italiane al Governo provvisorio libico, alla Repubblica di Gibuti, alla Repubblica del Pakistan ed al Governo dello Stato eritreo. Di particolare interesse vi sono inoltre le disposizioni che consentono alla Polizia di Stato di assumere personale, come agenti di polizia, utilizzando i posti vacanti del ruolo dei sovrintendenti e di prevedere procedure concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vicesovrintendente. Queste ultime norme sono volte a limitare gli effetti del blocco del *turnover* con positive ricadute in ordine al transito dei volontari dalle Forze armate nelle Forze di polizia. L'impegno italiano, come di consueto, si inquadra all'interno di missioni pienamente legittimate a livello internazionale, collocabili sotto l'egida delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza Atlantica; un impegno che testimonia l'importante ruolo svolto dal Paese a tutela della democrazia, della pace e della civiltà dei diritti umani e che costituisce un importante perno della politica estera. Esso deve pertanto essere sempre accuratamente ponderato in un costante e costruttivo dialogo tra Governo e Parlamento, anche perché la nuova legislatura presenterà delle sfide non meno impegnative di quella che si accinge a concludersi. Su tali basi, non posso che formulare, in qualità di Presidente della Commissione difesa, l'auspicio che alcune delle tematiche approfondite nella presente legislatura vengano riprese e concretizzate dal nuovo Governo e dal nuovo Parlamento. Mi riferisco, in particolare, alla necessità di introdurre una disciplina penale militare specifica a tutela del personale militare impegnato nelle operazioni di pace di mantenere un costante rapporto informativo tra l'Esecutivo ed il Parlamento, così che vi sia una costante valutazione delle singole missioni per razionalizzare al meglio le risorse economiche impiegate a favore di quelle maggiormente significative a livello internazionale. Signora Presidente, in conclusione, le preannuncio sin da ora il voto favorevole del mio Gruppo.

conosciamo le vicende che hanno condotto all'emanazione del decreto-legge di cui stiamo esaminando oggi in quest'Aula il provvedimento di conversione. La circostanza che fa sì che oggi siamo riuniti qui con le Camere *de facto* anticipatamente sciolte, non implica che certe importanti decisioni per il Paese vadano assunte frettolosamente, a cuor leggero e senza la discussione che meritano.

e, soprattutto, vanno fornite certezze ai nostri 6.000 militari di stanza all'estero in missioni internazionali di varia natura, quindi cercheremo di esporre la questione, come emersa a seguito dei lavori delle competenti Commissioni, in maniera sintetica, ma non per questo non esaustiva. In altre, diverse condizioni, con un Parlamento nella pienezza dei suoi poteri, avremmo potuto meglio confrontarci sul modello di presenza dell'Italia sulla scena internazionale, intanto facendo emergere le numerose perplessità che suscita in noi e potendo poi fare il punto sulle regole di ingaggio - tanto per fare un esempio tra quelli più stringenti - in caso di estensione della guerra civile siriana al Libano. In tale denegata ipotesi, infatti, UNIFIL 2 ci troverebbe (per non dire che troverebbe i nostri militari) impegnati nella polveriera mediorientale in maniera pericolosamente approssimativa. È vero, abbiamo il dovere di mettere al sicuro, attraverso il rifinanziamento delle missioni già in essere, i nostri connazionali. Ciò che proprio non emerge con sufficiente chiarezza da questo frettoloso e un po' abbondante, per quanto di altro vi è stato inserito, decreto decreto è la ragione per cui esso copra, in maniera del tutto originale, esclusivamente il periodo da gennaio a settembre 2013, lasciando invece scoperto l'ultimo trimestre dell'anno. Toccherà dunque al nuovo Governo trovare almeno altri 11 milioni di euro per la necessaria copertura. Si fa fatica a non intravedere un triste scaricabarile da parte del Governo Monti, quello, per intenderci, dei tecnici, dei professori. Altra anomalia del decreto oggi è in discussione è certamente la circostanza che in un decreto che reca nella intestazione la dicitura di «proroga delle missioni internazionali» si inseriscano ben 35 milioni di euro soltanto per le iniziative legate alla cooperazione. *Dulcis in fundo*, la parte del decreto che merita maggiore attenzione è quella che non costituisce affatto cooperazione allo sviluppo, ma una serie di disposizioni a esclusivo uso e consumo del Ministero degli affari

inviato all'estero (pubblici e privati) di essere collocati in aspettativa, nonché alle spese di viaggio per i congedi del personale, ma anche delle relative famiglie.

Si preferisce forse accontentare tutti, senza porsi troppe domande sulle strategie. Prendiamo il caso dell'Afghanistan. Finalmente, riportiamo a casa un terzo degli uomini. Lo facciamo però solo dopo che gli americani hanno fatto la stessa cosa, e per giunta dopo che altri Paesi europei hanno compiuto passi più radicali, come la Francia e l'Olanda, che hanno ritirato tutte le proprie truppe da combattimento. La lealtà all'America ed alla NATO sono certamente sacrosante, anche per noi della Lega Nord, ma non si capisce perché si debba sempre essere più realisti del re. A Washington sta prendendo quota il partito del ritiro completo dall'Afghanistan nel 2014, e forse prima. Auspichiamo di non essere proprio noi italiani quelli che ne prenderanno atto per ultimi. Nel frattempo, raccomandiamo ai nostri comandanti sul campo ed al Governo di essere prudenti e non far correre rischi inutili ai nostri ragazzi. Eventuali perdite oggi sarebbero infatti intollerabili, considerata la loro inutilità ai fini di una guerra e dell'intervento, che potrebbe anche incredibilmente concludersi con la completa riabilitazione dei talebani. Questi sono gli orientamenti che stanno infatti emergendo, anche se la nostra stampa ne parla poco o per niente. Anche in Libano manteniamo un contingente di 1.100 uomini in una missione ONU, l'UNIFIL 2, originariamente pensata per indebolire Hezbollah e separarlo dallo Stato ebraico. Nel frattempo, però, Hezbollah si è impadronito del Governo libanese e volge le proprie armi non contro Israele, ma contro gli insorti siriani. Verrebbe da chiedersi che senso abbia rimanere ancora nel Paese dei cedri, ma è un quesito al quale la contingenza non ci permette di rispondere. Comprendiamo bene, invece, e condividiamo pienamente la proroga delle missioni di contrasto alla pirateria marittima, la difesa della libertà di navigazione, specialmente quella di cui beneficiano i mercantili del nostro Paese, è sicuramente un interesse nazionale meritevole di tutela. Ma con una precisazione importante: occorre prudenza. E se vogliamo evitare altri incresciosi incidenti, come quello occorso ai nostri marò detenuti in India, è bene essere consapevoli dei limiti territoriali della nostra attività di contrasto alla pirateria, che deve focalizzarsi nelle acque antistanti la Somalia e non spingersi sino alle coste dell'India, qualsiasi forma assuma. Siamo lieti di osservare che la cooperazione con la Libia nel contrasto all'immigrazione clandestina è stata riattivata, anche se comprendiamo come sia inevitabilmente soggetta ai limiti imposti da una situazione obiettivamente difficile e conseguenza del disastroso intervento militare recente. Ci preoccupa invece l'espansione degli impegni militari terrestri nel Corno d'Africa e vorremmo capire qualcosa di più a proposito del rischieramento di 23 militari italiani nel Sahel, messi preventivamente a disposizione di un'eventuale missione europea per il Mali. Esattamente quanto sta accadendo in questi giorni ci ha spinto proprio questa mattina a chiedere al Governo qualche chiarimento in lo invitiamo a comunicare puntualmente e tempestivamente ogni evoluzione in quel teatro delicato. Vorremmo infatti sapere cosa cosa si pensa di fare e se per caso prenderà forza qualche penetrante e sostanziale assistenza all'eccessivo protagonismo delle truppe francesi, che siamo sicuri incontreranno non poche difficoltà nell'arginare l'espansione delle milizie islamiste a nord di Bamako. Non vorremmo pagare un nuovo, triste, tributo ad interventi non proprio bene coordinati, come quelli che ci hanno visto protagonisti nell'abbattimento del regime libico di Gheddafi. Vorrei attirare infine l'attenzione su due ulteriori punti. Il primo il provvedimento contempla anche cessioni a titolo gratuito di materiali militari a Paesi esteri. Roba vecchia, obsoleta, ai margini dell'inservibilità (almeno così si dice). Però a noi sembra lo stesso un azzardo regalare al Pakistan 500 blindati M113 per il trasporto truppe proprio mentre negoziamo con l'India il rilascio dei marò detenuti in Kerala. Islamabad e Delhi sono ai ferri corti, e non da oggi. Davvero non si poteva procrastinare questo dono? Il secondo punto è il nove mesi del 2013, rimettendo al prossimo Governo, che si insedierà dopo le elezioni, il compito di trovare i soldi per arrivare fino al 31 dicembre.

Siamo infatti consapevoli del fatto che è impossibile lasciare i nostri soldati privi delle necessarie garanzie economiche e giuridiche mentre rischiano la loro vita all'estero. Siamo grati a quei ragazzi e alle loro famiglie per quanto fanno e desideriamo ribadirlo in questa sede anche con il nostro atteggiamento. Vorremmo solo che si fosse più cauti nel modo in cui decidiamo della loro sorte. Non ci opporremo, quindi, alla conversione del decreto-legge

Questa affermazione, per quanto chiaramente comprensibile per certi versi, è il fallimento di quanto invece uno Stato membro di una unione politica dovrebbe perseguire, da una parte, e sicuramente un atteggiamento molto più vicino a politiche del secolo scorso piuttosto che a quelle che,

da consegnare ai libri di storia) gli obblighi internazionali di uno Stato membro delle Nazioni Unite piuttosto che esclusivamente l'interesse nazionale. questo perché siamo ormai al quinto giorno di un intervento militare deciso, indipendentemente da tutto ciò che la comunità internazionale stava costruendo, dalla Francia nei confronti di una sua ex colonia.

La Francia ha deciso di andare a bombardare un Paese, che per l'appunto è il vicino di un altro Paese che ha un problema simile, quello che lei, signora presidente Bonino,

la propria vita economica, civile e sociale - sicuramente non religiosa, perché non sono un gruppo fondamentalista - in un modo diverso da quello in cui, non solo dall'Ottocento ma sicuramente dal Trattato di Yalta in poi, si è invece andato dividendo il mondo. Questo Paese, che è vicino al Mali e fornisce la Francia dell'uranio necessario per le oltre quaranta Per evitare che il problema del Mali si trasferisse in Niger, dove sicuramente in parte già è presente, si è deciso di spostare l'attenzione mediatica internazionale con la scusa dell'impossibile creazione di una zona che non è sotto il controllo di nessuno e che è invasa - ho sentito dire più volte "occupata" - da gruppi terroristici. Ora, come un gruppo terroristico possa occupare

possano controllare alcunché. Quindi, si esagera un'emergenza e si creano le condizioni per intervenire esclusivamente con la mano militare piuttosto che con la politica.

che, all'epoca non ancora Ministro del Governo di transizione del Mali, era venuto in Europa principalmente per due questioni: innanzi tutto, per farci approfondire la conoscenza dello stato dell'arte del conflitto e, poi, per cercare sostegno

appello, sottoscritto da 1.300 personalità, di cui 300 parlamentari italiani, chiedeva una risposta pienamente politica ad un'emergenza che in parte era di sicurezza, ma in parte era anche

L'Organizzazione mondiale della sanità ha sviluppato studi e la Banca mondiale affronta da anni la questione dal punto di vista tecnico. Occorre, dunque, che il prossimo Governo si assuma una responsabilità politica molto chiara; probabilmente su questo tema, anche al di fuori delle Camere, i radicali saranno al fianco di chi farà prevalere il buon senso

sono chiamati ad affrontare insieme ogni anno, cioè la proroga delle missioni ed il loro relativo finanziamento. Desidero mettere in evidenza quanta importanza rivesta in questo contesto il ruolo svolto dalle nostre Forze armate, impegnate nelle azioni di contrasto al terrorismo ed anche nelle attività di polizia per il ristabilimento della legalità in quei territori. come tutto ciò si inquadri nel contesto di azioni finalizzate a garantire al nostro Paese sicurezza dentro e fuori i nostri confini, da parte di tutte le forze che appartengono a quel comparto sicurezza coordinato dalla legge n. 121 del 1981. In questi anni di stringenti riduzioni di politiche di bilancio, si mette in evidenza sempre più il rischio che la proiezione dell'efficacia dei compiti istituzionali si concretizzi in una diminuzione e in un arretramento della potenzialità delle nostre forze di sicurezza. Al riguardo, manifesto una preoccupazione e ne è prova

abbia anche deciso di finanziare solo i nove dodicesimi della partecipazione alle missioni internazionali. In tal modo si mette a rischio e a dura prova la capacità programmatoria verso la fine di quei mesi, non c'è dubbio, creerà un grande problema alla prosecuzione delle attività delle nostre Forze armate impegnate in quei teatri così complessi dove la programmazione delle risorse gioca un ruolo fondamentale.

il comma 5 dell'articolo 2 prevede un meccanismo positivo e favorevole per quanto riguarda le Forze di polizia.

all'attività di un Governo che noi abbiamo considerato in alcuni casi positiva e utile e in molti altri, invece, non positiva

al comparto sicurezza, così come in altre occasioni in passato, ma sempre di più e sempre meglio auspico, il grande valore che esso ricopre nel nostro Paese. In un momento in cui la domanda di sicurezza è crescente (e noi immaginiamo che possa crescere sempre di più), auspico che

la sicurezza del mondo così come per la sicurezza dell'Italia), si possa contare su forze di Polizia sufficientemente motivate

quel momento operava e non ha esitato a mettere a repentaglio la sua vita e la sua sicurezza per difendere quella di tutti noi. All'ispettore De Vincentis, che è stato ridotto in fin di vita da tre folli, da tre persone inqualificabili, pur non essendo in servizio, e che ha inteso difendere con il proprio impegno innanzitutto la divisa che portava e le istituzioni che rappresentava, va il mio pensiero e quello di tutti noi con l'augurio di una pronta guarigione ma, soprattutto, con l'auspicio

iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. In primo luogo, vorrei richiamare l'attenzione sulla copertura temporanea del presente decreto. È stato infatti rilevato da più senatori che la quasi totalità degli stanziamenti, a parte alcune voci, è relativa esclusivamente al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2013, coprendo quindi sostanzialmente solo i primi nove mesi di quest'anno. Ci sono alcune limitate e specifiche eccezioni. Tale scelta ha il lato positivo di realizzare una prospettiva coerente e di concreta continuità dell'azione portata avanti dal Governo e, al tempo stesso, di calibrare al meglio le decisioni che dovranno essere adottate dal prossimo Esecutivo.

che vede le forze internazionali ridurre progressivamente la propria presenza, con la parallela crescita della consistenza e delle capacità delle forze di sicurezza afghane. speriamo ovviamente ciò non avvenga), i mesi estivi in quel Paese sono comunemente definiti «la stagione dei combattimenti».

che, secondo quello che succederà la prossima estate, potremo avere un affinamento, una modulazione diversa della possibile prevista situazione di redistribuzione dei compiti alle forze afghane. In particolare, stiamo svolgendo un lavoro estremamente completo, aggiornato e coerente coi tempi previsti dalla nostra iniziare la riconsegna quasi totale delle cosiddette basi avanzate,

la difesa del proprio territorio. Speriamo che, coerentemente con la prospettiva data dalla comunità internazionale, in particolare dalla NATO, si possa riuscire a giungere al momento in cui dovremo fornire solo misure di assistenza tecnico-logistica e di addestramento ma non si svolgeranno più da parte nostra operazioni di combattimento, né si condurranno azioni di controterrorismo o di lotta al narcotraffico. Sulla base di questo calendario, già definito e approvato in sede internazionale, quindi, il nostro impegno ad uscire entro la fine del 2014 dalla presenza operativa in Afghanistan è mantenuto e confermato. Dirò di più: la forma e la consistenza dell'impegno italiano nel *post* ISAF saranno decise a tempo debito dal nuovo Governo e quindi prospettate al nuovo Parlamento. È tuttavia necessario identificare le più corrette modalità di ripiegamento del contingente nazionale,

Il successivo provvedimento di copertura degli ultimi mesi di quest'anno potrà, pertanto, recepire al meglio le esigenze operative che potranno nel frattempo emergere. Ciò detto, segnalo comunque come nel decreto in esame sia già stata prevista una consistente riduzione del nostro contingente in Afghanistan, il quale passerà dal livello medio di 4.000 militari mantenuto nel 2012 ad un livello medio di 3.100 militari nel corso dei primi nove mesi di quest'anno. In stretta aderenza con tale riduzione, diminuiscono anche le risorse assegnate a tale missione. Se nel corso del 2012 la partecipazione delle Forze armate alle missioni ISAF EUPOL in Afghanistan hanno assorbito un totale di 747 milioni di euro, nei primi nove mesi del 2013 il nuovo decreto include risorse pari a soli 426 milioni di euro. Per un raffronto più immediato, nel 2012 la spesa media mensile è stata pari a circa 62 milioni; nei la spesa media mensile sarà pari a 47 milioni circa. È doveroso da parte mia, a questo punto, introdurre il tema degli oneri specificamente connessi con la stipulazione dei contratti di assicurazione e trasporto associati alla permanenza dei nostri contingenti all'estero. Tali costi sono sempre presenti, per le ovvie necessità logistiche connesse con le missioni internazionali. Nel 2012, il totale di tali costi è stato pari a circa 140 milioni. Per Per l'intero anno 2013 - questa è una delle eccezioni di cui parlavo poc'anzi, per cui il riferimento è all'intero anno, e non ai primi nove mesi - lo stanziamento sarà pari a poco meno di 144 milioni di euro. Il lieve incremento è strettamente associato al ritiro di una grande quantità di mezzi e materiali dall'Afghanistan, ritiro che è ovviamente molto oneroso, ove si consideri la distanza di quel teatro operativo e la necessità di ricorrere ad una pluralità di vettori, aerei, navali e terrestri. La seconda delle missioni militari, per consistenza ed onerosità, inserita nel decreto è quella in Libano. In questo caso, non si prevede un significativo mutamento del nostro ruolo nel contesto della missione UNIFIL, né un cambiamento della consistenza del contingente, che rimarrà ad un livello medio di 1.100 militari, come nel 2012. La spesa per i primi nove mesi è pari a 118 milioni circa, ovvero in media di circa 13 milioni al mese, esattamente come nel 2012.

fra le diverse etnie e religioni, ma è stata anche di esempio e tutela per il rispetto dei diritti umani. Nei Balcani è invece possibile che la situazione sul terreno evolva per il meglio, con una fase di distensione e di pacificazione che consenta un'ulteriore riduzione della presenza militare internazionale. Ricordo come nel 2012 sia stato necessario dispiegare un contingente aggiuntivo di riserva, fornito per sei mesi anche dall'Italia. Per questo la consistenza media del nostro contingente, nel corso del 2012, è risultata pari a 848 militari, mentre nei primi nove mesi del 2013 la media sarà di 465, essendo terminato il dispiegamento della riserva. Il costo medio mensile del 2013 è quindi pari a 5,8 milioni, contro gli 8,2 milioni del 2012. Proseguendo con i contenuti del decreto, segnalo la continuazione delle operazioni antipirateria, condotte nell'Oceano indiano alternativamente sotto la bandiera dell'Unione europea o della NATO. L'impegno previsto è simile a quello dell'anno passato, con una presenza media di 237 militari (erano in media 261) e una

nella regione del Corno d'Africa e dell'Oceano Indiano. L'Italia partecipa infatti alla missione di addestramento delle forze somale (EUTM Somalia) e di sviluppo delle capacità marittime dei Paesi rivieraschi (EUCAP Nestor), ambedue sotto l'egida europea. La spesa associata a tali missioni è complessivamente pari a circa 7 milioni, nel periodo di copertura del decreto. Le altre attività all'estero delle nostre Forze armate proseguiranno senza significative variazioni. Segnalo comunque la novità rappresentata dal possibile prossimo avvio della missione a guida europea in Niger e Mali, come è stato ricordato in alcuni interventi, alla quale pensiamo di assegnare 24 militari, in media, nel corso dei nove mesi di copertura del decreto, per un importo complessivo di un milione e 900.000 euro. Per il Niger si tratta di una missione del tipo EUCAP di *capacity building* con la finalità di porre in atto l'organizzazione delle forze di sicurezza e di polizia. Per questa missione abbiamo già selezionato un uomo e prevediamo di poter partecipare con ulteriori otto unità. unità. Per il Mali, invece, si tratterebbe di una missione del tipo EUTM di *training assistance* a favore delle Forze armate maliane, basata su iniziativa dell'Unione europea in aderenza alle risoluzioni delle Nazioni Unite 2056, 2071 e 2085, per le quali pensiamo di fornire un contributo al massimo di 15 unità.

Segnalo inoltre che, a differenza del passato, il decreto 2013 prevede anche un finanziamento per l'impegno della Croce Rossa, in particolare con due medici e due infermieri in Afghanistan nonché con un medico e due infermieri negli Emirati Arabi, che in passato erano finanziati a parte. Complessivamente, quindi, il totale degli oneri inserito nel decreto per le missioni internazionali delle Forze armate è pari a 832 milioni di euro per i primi nove mesi del 2013. Per un più immediato raffronto con il 2012, evidenzio che corrispondono a 92,4 milioni di euro al mese in media - anche se, come detto, la rilevante voce dei trasporti in realtà copre tutto il 2013 - con una riduzione, rispetto alla media mensile dell'anno scorso, di 104,9 milioni di euro, molto prossima al 12

internazionali nei Balcani, in Nord Africa e in Afghanistan con contingenti ridotti, ma con un apporto importante. A questi interventi sono destinati circa 11 milioni di euro. Infine, alle attività di mantenimento del dispositivo informativo e operativo dell'AISE sono dedicati 10 milioni di euro. Il Governo, pertanto, tenendo fede agli impegni internazionali assunti dall'Italia e aderendo anche a nuove iniziative finalizzate al mantenimento della pace e della legalità internazionali, ha impostato questo tentativo di revisione dello sforzo da sostenere per le missioni internazionali, alla luce della prevedibile evoluzione della situazione nei terreni operativi, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza e gli interessi del Paese. l'azione del Governo cessa, lasciando un quadro di finanziamento che dovrebbe garantire, nei prossimi mesi, il rispetto degli impegni internazionali e la presenza del nostro Paese sul campo.

come esponente del Governo ci tenevo a ringraziare per il loro enorme contributo tutti i nostri connazionali, militari e civili, impegnati in queste importanti missioni internazionali. ai tre punti specifici. Avete insistito molto sul *timing* del finanziamento e sulla copertura per nove mesi. Credo che ci sia un eccesso di lettura

l'esigenza di una pianificazione a lungo termine con una flessibilità che in un certo modo corrisponde all'estrema volatilità della situazione in cui ci troviamo e che abbiamo discusso questa mattina in Commissione esteri; pertanto, non ci torno.

sottolineare, perché ci tengo a riconoscere il lavoro fatto dalla Commissione esteri del Senato quest'anno, che in realtà una parte degli stanziamenti è stata erogata direttamente attraverso la legge di stabilità sui fondi della legge n. 49 del 1987. Abbiamo avuto per la prima volta un grosso aumento, pari a circa 100 milioni di euro. Lo dico non solo per riconoscere che questo è anche il risultato dell'attenzione della Commissione esteri ai temi della cooperazione, così come il risultato del noto *Forum* di Milano del ministro Riccardi, ma anche per evidenziare che questa potrebbe essere una prima linea d'inversione di tendenza. Secondo me, quanto più il decreto sulle missioni, come strumento, comincerà a distinguere tra capitoli di spesa tanto meglio sarà. Quindi, nella parte del decreto missioni, secondo me, vanno i fondi di cooperazione effettivamente attinenti alle missioni internazionali (è stato detto da molti di voi), mentre va decisamente potenziato il capitolo «cooperazione bilaterale» attraverso la legge n. 49 del 1987. Infine vengo al terzo punto. Alcuni dei vostri interventi sembrano dire che a tratti

è evidente che siamo in una fase di disimpegno graduale che si completerà nel 2014. Emerge invece con tutta evidenza la salienza dei problemi di sicurezza per l'Italia particolarmente vicini nel Mediterraneo e in Africa. Su questo voglio dire soltanto una parola finale sul Mali.

alla politica europea, alle missioni europee e sul nostro contributo all'attuazione della risoluzione 2085 dell'ONU del dicembre scorso. È chiaro che il futuro Governo tornerà per discutere di questo in Parlamento.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo nel presupposto che: - con riferimento al comma 5, lettera *a)* dell'articolo 2,

siano rispettati i vincoli numerici e finanziari per le nuove assunzioni nel settore delle Forze armate e di pubblica sicurezza contenuti sia nell'articolo 66, del decreto-legge n. 112 del 2008 sia nei commi da 89 a 91 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013); con riguardo alla lettera *b)* del medesimo comma 5 dell'articolo 2, la decorrenza degli effetti giuridici ed economici connessi all'accesso alla qualifica di vicesovrintendente non abbia carattere retroattivo;

si rileva, tuttavia, che l'utilizzo di quota parte del fondo per le missioni internazionali di pace al fine di finanziare anche interventi di diversa natura non risulta del tutto conforme ai principi di corretta programmazione economica, oltre che alla legge di contabilità. In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta, fatta eccezione per la proposta 2.101, su cui il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

occupa la parte finale dell'articolo stesso, ai commi 30, 31 e 32, relativi alla dismissione del materiale, che per quanto ci riguarda presenta due ordini di problemi. Da una parte, come già evidenziato non soltanto da un'interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Turco alla Camera nell'agosto del 2009, ma da indagini indipendenti condotte sempre da parte del Partito per la tutela dei diritti di militari, gli M113 che noi daremmo alla Repubblica islamica del Pakistan potrebbero (ma siamo, con questo condizionale, più verso la sicurezza che verso l'insicurezza) essere contaminati da materiale radioattivo

essere accolta la notizia che il nostro Paese darà 500 veicoli M113 al Pakistan. Sicuramente i senatori presenti sapranno che stamani ci sono stati scontri a fuoco tra il Pakistan e l'India, in cui è morto un pakistano, nella solita regione del Kashmir. Sicuramente tutti i senatori presenti sapranno che la Corte suprema del Pakistan ha ordinato l'arresto del *Premier* pakistano per corruzione. Sicuramente tutti sapranno che il Pakistan è una Repubblica islamica che adotta

è probabilmente il primo Paese al mondo, assieme ai Paesi nordici, che quasi automaticamente concede l'asilo ai rifugiati eritrei. Noi, che abbiamo presentato pochissimi emendamenti, su questi tre riteniamo che occorra avere delle risposte da parte dei relatori e del Governo, perché in particolare per quanto riguarda i commi 31 e 32 ci sono problemi concatenati alla qualità del materiale dismesso e soprattutto alla qualità dei Paesi che vengono a prendere i soldi degli italiani.

Il tentativo di quest'ordine del giorno è di dare un significato politico alla nostra partecipazione alla missione ONU a Cipro, una delle più antiche missioni internazionali, tra l'altro una missione che dal 2004, cioè da quando l'isola è entrata nel territorio dell'Unione europea, si svolge appunto all'interno dell'Unione europea.

di continuare, certo, a porre in essere ogni utile azione sul piano delle relazioni bilaterali per consentire il dialogo tra la Repubblica di Cipro e la comunità turco-cipriota, ma chiediamo anche che il Governo, in contatto in contatto con i Paesi membri dell'Unione europea e i Paesi garanti di Cipro (la Turchia, la Gran Bretagna e la Grecia), porti avanti tutte le soluzioni per andare incontro alle due comunità. Tenga conto, signora che se è vero che Cipro fa parte dell'Unione europea, c'è una parte della popolazione a Cipro, quella turco-cipriota, che non fa parte dell'Unione europea, non ha gli stessi diritti degli europei, in quanto vive in condizioni di inferiorità per colpa di un blocco economico.

per aggiornare il mandato del contingente militare di stanza sull'isola facendolo evolvere da missione di pace a presenza di monitoraggio. si chiede al Governo di lavorare, sempre all'interno dell'Assemblea dell'ONU, per il riconoscimento di un particolare *status* per l'Entità turco-cipriota sulla base di quanto recentemente fatto per la Palestina. Non voglio entrare nel merito della scelta del Governo che ha di fatto riconosciuto lo Stato palestinese, ma indubbiamente questo rappresenta un precedente che in situazioni non del tutto similari, ma comunque in situazioni che presentano alcuni aspetti similari, non può essere ignorato. Non so cosa vorrà dire il Governo su questo punto; io sono convinto comunque che senza un riconoscimento anche alla comunità turco-cipriota non arriveremo mai ad

europea; l'altra, la parte turco-cipriota, non ha avuto nulla, e secondo me, se non le si va incontro con qualche forma di riconoscimento, continuerà a non avere nulla e il problema annoso di Cipro continuerà a tormentare gli europei e l'Unione europea. *(Applausi del

avanzate dal senatore Perduca circa le condizioni di pericolosità radioattiva o meno dei materiali

continuare a prevedere il rapporto e il confronto quadrimestrale tra Governo e Commissioni affari esteri e difesa del Senato e della Camera sugli argomenti che stiamo trattando oggi.

M113 senza armamenti e in uno stato di degrado. La cessione comunque si inquadra nell'ambito di un *memorandum* d'intesa

il futuro della comunità turco-cipriota e della pacificazione a Cipro, proporrei una riformulazione, partendo dalla nostra convinzione che il parallelo fra Cipro e la Palestina non sia opportuno. In sostanza, propongo di togliere,

senatori, siamo vicini a questa vostra sensibilità politica; riteniamo tuttavia che lo sforzo internazionale su Cipro, che voi del resto ricordate nelle premesse, è volto a rendere possibile un'unificazione pacifica con una comunità binazionale e federale, mentre nel caso della Palestina la soluzione indicata da tutti, anche da chi ha votato contro all'ONU, è la formula dei due Stati.

Tra l'altro, ricordo che il semestre conclusosi il 31 dicembre vedeva presidente di turno la Repubblica di Cipro ricevere il premio Nobel per la pace, con rispetto parlando, da parte del comitato Nobel. In secondo luogo, è vero: non c'è niente a che vedere tra l'Autorità nazionale palestinese

la voglia di distruggere lo Stato con il quale si ritiene non si debbano mai unire solo perché si tratta di una democrazia.

non è parsa particolarmente convincente la risposta del sottosegretario Magri ai rilievi

che ha un conflitto in corso con un Paese con il quale abbiamo un contenzioso aperto, per due responsabili di un atto ancora tutto da verificare, che fanno riferimento al Ministero della difesa. Comprendendo sicuramente gli accordi pregressi, occorre essere molto cauti.

sono passati alla storia proprio per essere anch'essi un'ulteriore tentacolo di un regime totalitario. Torno a ripetere che noi prima regaliamo veicoli al Pakistan e adesso all'Eritrea, Stato dittatoriale dal

criminali, devono eventualmente essere portati davanti ad una corte e non morire per malattie da noi causate, per le quali magari saremmo anche coinvolti in un altro tipo di cause internazionali. Chiedo pertanto anche per questo

G2.100 e G2.101, in quanto estranei all'oggetto della discussione. L'emendamento 2.101 reca infatti disposizioni, di natura ordinamentale, relative allo sviluppo della carriera degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri; allo stesso oggetto si riferisce altresì l'ordine del giorno G2.101. L'ordine del giorno G2.100 attiene invece ai profili finanziari relativi alla revisione dello strumento militare nazionale.

questo è quasi sicuramente l'ultimo intervento che chi vi parla svolge nell'Aula del Senato.

dei nostri militari e degli interventi di sostegno, cooperazione e ricostruzione nei Paesi in cui queste missioni si svolgono, proprio perché è uno di quei provvedimenti su cui

alla Camera dei deputati, hanno avuto l'occasione non soltanto di esprimere il proprio consenso, ma - come chi vi parla - di contribuire in molte circostanze alla redazione dei testi di questi provvedimenti (che arrivano

trasferimento alle competenti autorità di polizia e di sicurezza afghane della sicurezza dell'Afghanistan, ma questo è e sarà possibile solo grazie all'opera svolta in tutti questi anni, dai nostri soldati, dagli appartenenti alle Forze armate. Nei giorni Nei giorni scorsi abbiamo salutato, a Solbiate Olona, la partenza dello *staff*, di tutta l'organizzazione del Comando di proiezione rapida della NATO, comandato dal generale Battisti, che si schiererà

significativo e mai da sottacere è l'impegno della UNIFIL che, sotto la guida del generale Serra, continua a svolgere egregiamente una funzione di interposizione, mantenimento e ristabilimento della pace nello scenario libanese.

la partecipazione alle missioni nell'Oceano Indiano, sia quella sotto l'egida UE, *Atalanta*, sia quella sotto l'egida NATO, *Ocean Shield*

francamente, di quanto è stato finora, perché finalmente questa vicenda veda la fine con il rientro definitivo dei nostri due sottufficiali del San Marco ancora detenuti illegalmente in quel Paese. Tutte le altre missioni, circa 15, che sono ancora una volta prorogate, pur con un numero di unità molto ridotto, hanno un'importanza decisiva, fondamentale non solo per la sorte dei Paesi dove i nostri contingenti sono schierati ma specialmente perché attraverso l'azione dei militari e dei civili che partecipano a tali missioni si svolge la gran parte della politica estera italiana. Non possiamo dimenticare, e il Parlamento deve in ogni caso ricordare, che si si tratta della principale forma di presenza dell'Italia sullo scenario internazionale che è, peraltro, corroborata dalla partecipazione elevatissima fra i maggiori Paesi contributori sia in termini militari che in termini economici. Noi, nel rinnovare questo grande apprezzamento, dobbiamo anche rilevare, come ha fatto egregiamente il senatore del nostro Gruppo Alfredo Mantica, intervenendo in sede di discussione generale dall'alto della sua grande esperienza pluriennale come Sottosegretario

non ci convincono: non ci convince la strana durata di nove mesi, che non coincide né con i sei né con i dodici del passato e non coincide con la fine dell'opera del Governo attuale di questa legislatura, e quindi ci è sembrata un temporizzazione

gli stanziamenti per la ricostruzione e la stabilizzazione in aree di forte criticità come la Siria, con le incongruenze riferite allo stesso Parlamento siriano, (non si sa bene quale se l'attuale e il futuro), o alle vicende altrettanto singolari, in termini di determinazioni,

nostra grande volontà di continuare a partecipare a queste missioni. I senatori del Gruppo Fratelli d'Italia-Centrodestra Nazionale, con il proprio voto favorevole a questo provvedimento, confermano la coerenza e la linearità di tutti i voti che hanno espresso nelle similari occasioni passate. Specialmente però riaffermano con forza il sostegno, la profonda gratitudine

Prima di affrontare nel merito il provvedimento al nostro esame, vorrei solo ribadire come, a prescindere dall'esito delle future elezioni, non posso che essere soddisfatta e orgogliosa del lavoro svolto durante questa legislatura dal Gruppo dell'Italia dei Valori qui al Senato. Tornando all'oggetto del mio intervento, come già è stato anticipato stamane dal collega Caforio, devo subito ribadire che il Gruppo dell'Italia dei Valori,

è stata chiara e netta da sempre, sin dall'inizio di questa legislatura. Abbiamo, infatti, dimostrato il nostro favore con riguardo alle sole missioni internazionali di pace in senso stretto. Le numerose missioni internazionali portate avanti dai nostri soldati mi riferisco a quelle veramente di pace, come quelle nel Libano, nei Balcani e nel Medio Oriente - indubbiamente rappresentano il fiore all'occhiello della nostra attività internazionale. Tuttavia, questo Governo, uniformandosi purtroppo a quello che lo ha preceduto, ha deciso di non rivedere la posizione dell'Italia sulla missione in Afghanistan, come in passato sull'Iraq. Secondo quanto previsto dal decreto-legge in titolo infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, si autorizza la spesa di 426 milioni di euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni ISAF e EUPOL in Afghanistan. In proposito, colleghi, non posso non sottolineare che sono ormai trascorsi ben dieci anni dalla nostra presenza in quella Regione e che i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I talebani sono sempre più forti, il traffico di droga è aumentato, i signori della guerra si sono arricchiti, la corruzione regna sovrana, le elezioni, secondo quanto certificato da organismi internazionali, sono state inficiate da brogli di ogni genere e le donne, e soprattutto i bambini, vivono una situazione di pericolo costante. È evidente ormai che la missione di pace alla quale era stato destinato il nostro contingente ha prodotto un fallimento. È altrettanto evidente che tale missione nel corso del tempo ha cambiato la propria natura trasformandosi in presenza militare, in violazione dell'articolo 11 della nostra Costituzione. A conferma di quanto appena affermato, basti ricordare che per le sole missioni ISAF e EUPOL il nostro Governo ha stanziato dal 2002 ad oggi oltre 4 miliardi e mezzo di euro, dei quali circa il 90 per cento è stato destinato per armamenti ed equipaggiamento e solo il restante dieci per cento per interventi di carattere civile, di ricostruzione e aiuto alle popolazioni. Per questi motivi riteniamo che i nostri ragazzi - così molto spesso li chiamiamo in quest'Aula - tornino a casa, perché non possono continuare a combattere una guerra non loro sotto il falso vessillo della missione di pace. Ci dispiace ovviamente di dover votare contro anche il rifinanziamento delle altre missioni di pace e contro i contributi finanziari per la cooperazione allo sviluppo, fra l'altro ancora una volta non sufficienti. Tuttavia, non ci è possibile cambiare posizione, a causa dell'ostinazione dei governi a ritenere quella afghana una missione di pace. Signor Presidente, colleghi, concludo raccomandando a coloro che tra poco si troveranno a dover portare avanti il lavoro fin qui svolto di tenere sempre presente, nell'assicurare il sostegno alle missioni internazionali, l'ormai noto articolo 11 della nostra Carta costituzionale. Ringraziando tutti per l'attenzione, anche se oggi un po' scadente, e per la disponibilità che mi avete sempre riservato, dichiaro quindi il voto contrario del Gruppo Italia dei Valori sul disegno di legge di conversione del decreto-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali.

il voto ovviamente favorevole del mio Gruppo, nonostante alcune perplessità personali, relative ad un emendamento che ho ritirato su richiesta dei relatori, che riguardano non tanto la parte militare del provvedimento, quanto la cooperazione internazionale,

in particolare in Afghanistan, nei Balcani e in Libano, dove si è riusciti, attraverso i nostri soldati, la nostra difesa, attraverso gli uomini che ci rappresentano in tutto il mondo, ad essere presenti e a discutere nei tavoli internazionali con Stati Uniti Stati Uniti e Gran Bretagna ad un livello alto e importante, cosa che forse prima sinceramente mancava. Siamo riusciti a tenere questo ruolo nonostante i tanti presenti problemi all'interno del nostro Paese. La bandiera quindi è stata tenuta alta, oltre che dai nostri civili che lavorano per gli organismi internazionali e non solo, anche e soprattutto dai nostri uomini

Grazie, potrà dare più sicurezza e più forza a quello che di fatto è il bene comune che il militare fa non solo ed unicamente

infatti, operano professionisti di tutti gli ordini (dottori, ingegneri, architetti) capaci di costruire ponti, città, strade,

sarebbe importante - e mi rivolgo a lei, signor Sottosegretario - che venisse apprezzato anche quello che ha fatto il nostro partito, che - come lei sa benissimo - è in una condizione diversa dagli altri: siamo stati fuori dal Governo, non abbiamo condiviso niente; l'unica materia che abbiamo condiviso, e su cui abbiamo lavorato

innovativo per quello che riguarda la nuova situazione che si andrà a creare per il settore militare - lei sa benissimo che in più modi ho cercato di spiegarvi che le cose andavano fatte in un certo modo.

mio avviso delle volte in maniera anche abbastanza grottesca, perché quando si decide di fare una cosa la si deve fare fino in fondo. La riforma dovevamo farla meglio, non l'abbiamo fatta, e comunque non l'abbiamo fatta aiutando i militari.

e probabilmente non si è riusciti a fare di meglio. Noi, per senso di responsabilità, come ho evidenziato anche in Commissione, votiamo a favore, per cui non ci sottraiamo alla lealtà nei confronti soprattutto dei militari e del settore.

bene o male siamo riusciti a darci una logica di ragionamento in Commissione, e anche per questo volevo ringraziare tutti i commissari che hanno operato in questa legislatura e che hanno lavorato tutti, chi più chi meno, con una certa saggezza, con una certa solerzia e capacità.

Però, questo non ci fa non pensare che è stata una testimonianza (l'ho detto anche oggi), tutto sommato, di bontà del Parlamento.

ma con decoro, perché sono l'unica situazione che dà luce alla politica estera del nostro Paese. Però non si può essere i gendarmi del mondo, l'ho detto anche l'altra volta: dobbiamo stare con decoro nelle missioni nelle quali possiamo

della Libia. Con il Mali bisogna stare attenti. Parliamo di zone in cui c'è una cultura tribale che non è la nostra.

voterà a favore del decreto sulle missioni internazionali e sui progetti di cooperazione internazionale. Lo farà seguendo una tradizione ormai consolidata nel ormai consolidata nel corso delle ultime legislature, in particolare in questa. Anche dall'opposizione non abbiamo mai fatto mancare il nostro voto di consenso alle missioni, non solo per il giusto, doveroso omaggio e riconoscimento al prezioso lavoro che compie il nostro personale militare e civile in giro per il mondo, ma perché condividiamo nel fondamento l'idea stessa di una proiezione del nostro Paese a livello internazionale anche attraverso l'uso legittimo e misurato della forza. L'articolo 11 della Costituzione impegna l'Italia a ripudiare la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, ma poi aggiunge che l'Italia opera in maniera fattiva per costruire un ordine internazionale fondato sulla giustizia e sulla pace tra le Nazioni. Quindi, il pacifismo - per così dire - della Repubblica italiana non è neutralismo o isolazionismo, bensì una forma di interventismo attraverso il multilateralismo delle istituzioni internazionali. Da questo punto di vista abbiamo esercitato sempre una funzione di attenzione critica come Gruppo parlamentare nei confronti dei Governi sia quando siamo stati maggioranza sia quando siamo stati all'opposizione, perché abbiamo sempre sottolineato tre punti fondamentali che ci sono sempre stati molto a cuore: il primo è l'assoluto rispetto della legalità internazionale. L'uso legittimo della forza nelle situazioni di *peace keeping* o anche di *peace enforcing* - come in alcuni casi è accaduto - è tale, cioè legittimo e quindi anche utile ai fini della costruzione della pace, se nel deciderlo si segue la via, spesso faticosa e lunga, a volte anche non priva di difficoltà, della legalità internazionale e delle istituzioni internazionali, a cominciare dalle Nazioni Unite. Esemplare è il caso recente della Libia, dove siamo potuti intervenire - come era giusto e doveroso fare - soltanto a seguito dell'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

progressivamente aggravando e incancrenendo anche perché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha trovato il consenso per autorizzare una qualche forma di uso della forza, sempre misurata, proporzionata e legittima. Questo è stato il primo punto di riferimento che abbiamo sempre seguito: abbiamo detto no a missioni che fossero al di fuori della legalità internazionale, come è stato, dal nostro punto di vista, l'intervento americano in Iraq; abbiamo invece sempre detto di sì convintamente alle missioni all'interno dell'alveo della legalità internazionale. Il secondo punto che abbiamo sempre seguito è quello di un riequilibrio, per quanto possibile, tra le risorse stanziate per gli interventi di carattere militare e quelle stanziate per la cooperazione civile. Sotto questo profilo non possiamo non rilevare con soddisfazione che il Governo Monti ha segnato un'inversione di tendenza significativa, che ha premiato i nostri sforzi.

Bisogna fare di più e di meglio per la cooperazione; è una delle cose che questa legislatura trasmette alla prossima - insieme ahimè per l'ennesima volta - all'insuccesso

un testo approvato dalla Commissione, che trasmetteremo al prossimo Parlamento). Infine, il terzo punto che abbiamo sempre perseguito è quello del metodo, in particolare

Sotto tale profilo dobbiamo registrare una battuta d'arresto. Questa volta il decreto avrà vigenza solo per nove mesi. Siamo naturalmente in una fase di cambio di legislatura, per cui non ci sentiamo di condividere critiche a mio modo di vedere - che hanno fatto altri Gruppi. Certamente il decreto annuale è una buona tradizione da

Siamo di fronte ad un passaggio importantissimo. Questa è la politica con la "p" maiuscola, la politica che decide della proiezione internazionale di un Paese e dell'uso della forza. Non esiste niente di più delicato

È intuibile che ciò sia dovuto alla necessità di controllare la disponibilità del bilancio dello Stato per tale settore. Questo, però, non può evitare anche un'altra constatazione: purtroppo la ristrettezza eventuale di bilancio cade in un periodo di cambiamento di molti aspetti tradizionali delle missioni internazionali.

viene letta la capacità di un Paese di far fronte responsabilmente alle sfida di stabilità e sicurezza che la comunità internazionale è chiamata a fronteggiare.

NATO. Proprio in tale ambito vedo un secondo cambiamento, ossia un mutamento della strategia della NATO nel contesto della sua presenza nelle varie situazioni internazionali: una presenza sempre più orientata alle attività di formazione e assistenza alle forze di sicurezza nazionali. Si tratta di interventi che assicurano una cooperazione più accentuata allo sviluppo e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. È probabilmente questo l'inizio di un cambiamento ragionato che tiene conto anche delle situazioni nuove che, come è stato più volte ricordato da colleghi proprio stasera, si prospettano nei vari Paesi. per queste forme di presenza che stanno gradatamente prendendo consistenza, personalmente auspico che la politica estera - anche quella del nostro Paese - assuma una consistenza che superi la semplice presenza delle Forze armate. Credo che la presenza, anche geografica, del nostro Paese dia la possibilità di partecipare a questa evoluzione dei rapporti internazionali e della presenza di organizzazioni internazionali. Oltre a ciò, ritengo che l'evoluzione ed il cambiamento che stanno caratterizzando molti Paesi siano la conseguenza di uno sforzo che dobbiamo interpretare nel modo più ampio.

la caratteristica fondamentale della nostra politica estera al Ministero della difesa. Lo sottolineo con tutto il rispetto per il Ministro della difesa, il Dicastero tutto e gli italiani che vanno

l'uso legittimo e misurato della forza, e questa è una nostra caratteristica all'interno dello scenario internazionale per quanto riguarda le organizzazioni internazionali o regionali. Tuttavia non posso accettare, da parte di un rappresentante di uno dei più grandi partiti politici italiani, la menzione del rispetto della legalità internazionale quando in Italia quotidianamente si calpesta la legalità costituzionale.

dell'attività di gestione dei rifiuti urbani nella Regione Campania che, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 95, del 6 luglio 2012 viene prorogata con le stesse modalità fino al 30 giugno 2013. Anche il termine per il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore a 13.000 kJ/kg

anche sugli argomenti che ha trattato la Commissione. Sono stati infatti approvati in Commissione alcuni importanti provvedimenti, sempre con l'obiettivo di spostare dei termini o di intervenire su situazioni emergenziali nazionali di grande rilievo (come il terremoto in Emilia), che hanno già catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica.

la sua risoluzione conclusiva relativa all'indagine conoscitiva sulla gestione del trattamento dei rifiuti e sui costi nell'intero territorio nazionale. Nel ringraziare tutti i componenti della Commissione che hanno partecipato ai lavori di tale indagine, ed in particolare la senatrice Mazzuconi che ne è stata la relatrice, debbo evidenziare come le relative conclusioni, oltre a toccare tutta una serie di criticità che sono ancora presenti sull'intero territorio nazionale soprattutto riguardo alla disomogeneità normativa che presiede al fenomeno della trattazione dei rifiuti, che quindi richiederebbe un'impellente normativa quadro per ricondurlo quanto meno nelle linee generali e complessive, nell'ambito di norme certe e applicabili su tutto il territorio nazionale,

tassa, che dovrebbe essere correlata ai servizi e quindi essere una tariffa (non una tassa) e in quanto tale non dovrebbe esorbitare oltre il costo sul cittadino dello svolgimento del servizio, è stata inopinatamente trasformata in una patrimoniale, perché riguarda le consistenze degli immobili piuttosto che gli gli abitanti degli stessi e il quantitativo dei rifiuti prodotti. In tal modo si rischia un duplice effetto: la non correlazione tra l'incidenza dell'attività del cittadino

altro Comune, che si troverebbe a pagare questa tassa per tutto l'anno e non solamente per il periodo in cui gode del servizio corrisposto. Così come manca completamente la correlazione tra rifiuto prodotto e consistenza dell'immobile e del nucleo familiare. Tutte queste criticità sono sottolineate nella relazione approvata dalla Commissione e hanno spinto la stessa ad interrogarsi sulla opportunità di differire il termine di attivazione della TARES, non tanto dal punto di vista della competenza, quanto e soprattutto dal punto di vista della cassa. Vi è infatti anche un motivo politico forte su questo, Presidente e colleghi: ad aprile, quando sarebbe prevista l'esazione della prima rata non ci sarà ancora il nuovo Governo, quindi, nessuno avrà avuto la possibilità eventualmente di incidere sulla TARES, secondo le sue propensioni

la Commissione ha ritenuto di dover approvare un emendamento che differisce al 1° luglio l'entrata in vigore della TARES,

Un Governo che dovesse infatti insediarsi ai primi di aprile, così come previsto nel nostro calendario politico-parlamentare, avrebbe tutto il tempo eventualmente per adottare, in termini di urgenza ma anche di pacata discussione parlamentare, un provvedimento utile a diminuire l'incidenza della TARES sui bilanci familiari e soprattutto restituire alla TARES la sua natura di tariffa per un servizio corrisposto,

Il Governo in Commissione bilancio ha chiesto che questo provvedimento venisse coperto, come si dice in termine tecnico, con cospicue somme, e ha fatto due operazioni che rivelano che rivelano la natura vera di questa tariffa TARES. In primo luogo, ha riconosciuto che non vi è una correlazione tra il servizio e l'imposta, perché se così fosse non ci sarebbe bisogno di nessuna copertura una imposta che esorbita il costo del servizio e quindi crea un introito alle casse dello Stato e degli enti locali che non trova una corrispondenza nel costo del servizio.

vessatorio nei confronti delle famiglie e delle imprese perché questa è la politica che ha impresso anche nell'attuazione dei decreti attuativi dell'IMU e di altre corrispondenti imposte.

giorno e minuto in cui saremo costituiti in Assemblea parlamentare dobbiamo difendere e sostenere gli interessi di 60 milioni di italiani riteniamo che ci debba essere la possibilità di uscire dal vincolo di questa TARES impropria, e ciò può accadere naturalmente - cosa che condividiamo - solamente con un Governo politico nuovo, ammesso che questo ormai non sia anche un Governo politico, che possa prendere le sue determinazioni, d'intesa anche con gli enti locali, come uno dei suoi primi atti. È chiaro che ognuno auspica di poter essere al Governo e ognuno ha le sue ricette per ovviare a questa improprietà di una tariffa diventata tassa. Debbo sottolineare ancora una volta, ad onore dell'intera Commissione, che la mia proposta emendativa è stata votata

il Governo nella sua rigida interpretazione o nel mantenimento della sua volontà originaria, per addivenire comunque ad un differimento del pagamento della prima rata della TARES 2013 a luglio, in maniera, ripeto, tale da consentire al nuovo Governo di adottare un eventuale intervento lenitivo di questo balzello, che va ad aggiungersi impropriamente ad altri già estremamente pesanti sul bilancio di famiglie e imprese.

di modificare i parametri quantitativi e percentuali di intervento sulla ricostruzione. In tal modo, si potrebbe superare una situazione di fatto che mi dicono si sia creata in Emilia:

di contributo rispetto al costo sostenuto e di poter utilizzare effettivamente una norma che questo Parlamento ha varato cercando di venire incontro alle esigenze delle popolazioni terremotate.

Grazie,

Questo provvedimento, ripeto, risolverebbe tantissimi problemi, anche perché l'ultima direttiva comunitaria in tema di rifiuti ci indica la strada della semplificazione

nei confronti dei cittadini, autorizzando l'approvazione di questa norma. Ho illustrato le tre questioni sulle quali la Commissione si è intrattenuta. Ancora una volta non posso non ringraziare tutti i componenti della Commissione

nonostante la vicinanza delle elezioni, ancora una volta la Commissione ambiente e l'intero Parlamento abbiano dato un segnale di assoluta coerenza con il mandato a suo tempo ricevuto dai cittadini.

il decreto-legge ambientale del ministro Clini costituisce probabilmente l'ultimo atto di questa legislatura. Rappresenta dunque un buon momento per un bilancio ambientale del Governo Monti e dell'intero quinquennio. Un bilancio francamente deludente: deludente l'attenzione dedicata all'ambiente, deludenti le risorse ad esso destinate. Sono state perse occasioni importanti per aggiornare la normativa contro gli inquinatori e i danni ambientali, si è colpevolmente tralasciato - pur avendo l'occasione del termine di recepimento della direttiva quadro - di inserire i delitti ambientali nel codice penale, come invece richiesto da ampia parte degli esperti, della dottrina e della giurisprudenza. Abbiamo facilitato trivellazioni e perforazioni petrolifere inutili se non dannose, abbiamo semplificato alcune procedure per le rocce da scavo, ma il bilancio resta marcato dalla sanatoria concessa all'impianto ILVA, di cui dovrà presto occuparsi la Corte costituzionale. In materia di consumo di suolo tutto si conclude con un nulla di fatto, mentre solo per l'assetto idrogeologico possiamo sperare, se non nel necessario intervento sulle competenze, almeno in una riorganizzazione del coordinamento nazionale. Per l'efficienza energetica siamo lontani da una stabilizzazione degli incentivi, mentre per il settore del fotovoltaico e del solare si è vissuto un vero e proprio biennio di assedio. Per il resto, abbiamo visto soprattutto deroghe e proroghe come quelle contenute in questo modesto decreto, il primo e l'ultimo del 2013. Nella Regione Campania è in vigore dal 2010 un regime "temporaneo" per cui spettano alle Province le funzioni di gestione per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti urbani. Ai Comuni, invece, spettano solo (la parola "solo" è menzionata dall'articolo 11) le funzioni di raccolta, spezzamento e trasporto, oltre a quelle di smaltimento o recupero dei rifiuti della raccolta differenziata. La legge prevedeva il passaggio dal regime speciale delle competenze a quello ordinario a partire dal 1° gennaio 2013. Due settimane dopo questa data, e con la motivazione che non si vuole che il passaggio aggravi le criticità esistenti o ne crei di nuove, si introduce una norma transitoria che prolunga fino al 30 giugno 2013 il regime speciale. Solo dal 1° luglio, quindi, ai Comuni tornerà l'organizzazione e la gestione dei servizi concernenti i rifiuti urbani, con la riscossione dei relativi tributi. Già nel 2010, inspiegabilmente, invece, non si era voluta accogliere una proposta emendativa di assoluto buonsenso, con la quale si chiedeva di non esautorare dai propri compiti e competenze i Comuni campani che hanno sempre rispettato, raggiunto e superato i livelli di raccolta differenziata e gli *standard* di gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, a beneficio di società provinciali che moltiplicano i costi e non hanno la consolidata esperienza sul campo. Vengono, quindi, penalizzati Comuni virtuosi, parificandoli a quelli inadempienti. Si tratta di una misura irragionevole e contraddittoria rispetto alle finalità del superamento dell'emergenza. L'articolo 1, comma 2, proroga di un ulteriore anno l'entrata in vigore di un divieto sancito addirittura nel 2003, relativo allo smaltimento in discarica dei rifiuti con un determinato potere calorifico. L'entrata in vigore di tale divieto, contenuto nel decreto legislativo n. 36 del 2003, era stata più volte prorogata fino al termine del 31 dicembre 2012; è sempre stata fatta slittare con la motivazione che in Italia non sono presenti strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un potere calorifico come quello indicato nella norma. Vuol dire che da dieci anni abbiamo una disposizione nell'ordinamento che non è mai entrata in vigore. Ciò significa averla tacitamente abrogata. È francamente sconcertante che per importanti settori industriali produttivi del Paese, quali, ad esempio, l'industria alimentare, cartaria, tessile, fino ad oggi, per effetto di ripetute proroghe dell'entrata in vigore della norma, la discarica ha rappresentato la sola soluzione praticabile. L'articolo 2, a sua volta, costituisce una deroga ad un principio generale da poco stabilito. Il Governo ha voluto dapprima decidere la non reiterabilità delle gestioni commissariali ambientali; poi si è reso conto che tale disposizione avrebbe causato pericolosi vuoti di attività per il superamento di alcune emergenze. Pertanto, ci si è limitati ad una proroga circoscritta alla bonifica di Giugliano e dei laghetti di Castelvolturno, allo stabilimento Stoppani nei Comuni di Arenzano e Cogoleto e al naufragio della nave Concordia, i cui lavori di messa in sicurezza e rimozione continuano a slittare ad un anno e tre giorni dal momento della tragedia davanti all'Isola del Giglio. È trascorso un anno dal disastro della Costa Concordia, ma il relitto è fermo all'Isola del Giglio e resterà lì ancora per mesi. Se da un lato appare necessario mantenere lo stato d'emergenza per favorire il recupero e il trasferimento della nave, dall'altro non si può tacere che in questo anno è stato fatto molto poco. Il cronoprogramma aggiornato delle operazioni prevede la rimozione del relitto entro la fine dell'estate 2013, ma è già stato annunciato l'ennesimo ritardo che farà slittare la conclusione degli interventi a dopo settembre 2013. La Costa Crociere ha dichiarato, proprio nei giorni scorsi, che sarebbe addirittura fuorviante e poco attendibile determinare una data esatta. Noi, invece, non possiamo che chiedere di accelerare i tempi di rimozione del relitto, così da ripristinare al più presto l'ecosistema marino. I continui ritardi non fanno altro che aumentare il rischio di nuovi e pericolosi sversamenti in mare di sostanze tossiche presenti nel corpo galleggiante. I ripetuti slittamenti nei tempi dei lavori di messa in galleggiamento e rimozione necessitano quindi di spiegazioni precise, spiegazioni che vi avevamo già chiesto con un'interrogazione presentata nel mese di luglio dello scorso anno, in cui veniva sottolineato come, di fronte ad una tale emergenza ambientale, qual è quella che si è verificata a ridosso della costa gigliese, non si sia attentamente vigilato sulla necessaria trasparenza delle procedure, lasciando la quasi totale libertà all'armatore nella scelta del migliore percorso da seguire per la rimozione della nave. Siamo convinti, dunque, che, al di là della proroga dei poteri emergenziali, occorra a questo punto sottoporre il progetto prescelto ad una attenta revisione per evitare di dilazionare ulteriormente i tempi, considerato anche l'aumento esorbitante dei costi di intervento (oltre il 25 per cento) che supera i 400 milioni di dollari. Tale incremento, unito alle continue modifiche e variazioni del progetto, è una dimostrazione più che evidente della debolezza degli interventi programmati. Il ritardo accumulato - è evidente - ha le sue motivazioni tecniche ma resta innegabile. Anche su questo, come sul complesso delle politiche ambientali, non resta che sperare in un deciso cambio di marcia della nuova legislatura, in cui difesa del suolo, *green economy* e crescita abbiano ben altre prospettive di quelle esplorate negli ultimi cinque anni.

il terremoto è avvenuto alla fine di maggio e nelle zone terremotate non è ancora stato speso un euro di denaro pubblico per quanto riguarda la ricostruzione. Soltanto l'11 gennaio il dottor il dottor Befera ha adottato un provvedimento per cercare di chiarire il famoso articolo 3-*bis* sul credito di imposta in capo ai beneficiari, che può essere messo esclusivamente in compensazione delle rate degli interessi. Sulla base di tale provvedimento, poi, le singole banche dovranno andare a firmare con la Cassa depositi e prestiti delle convenzioni in virtù delle quali saranno in grado, in un prossimo futuro, di erogare dei mutui. Faccio presente che sono passati

o convocato i parlamentari dell'Emilia-Romagna per fare una valutazione sul terremoto. Ha però sfornato decine e decine di ordinanze, in una delle quali ha scritto che il massimo del contributo che si può avere sui famosi sei miliardi della Cassa depositi e prestiti è

fino all'80 per cento di quella quota parte. E il resto chi glielo dà? Chi è che concede loro il finanziamento per poter completare il lavoro? Siamo ancora alla completa paralisi, rispetto alle procedure che non sono state ancora completate per permettere di accedere ai mutui, sia per questa totale incertezza sul *quantum* che coloro che hanno subito danni dal terremoto potranno percepire.

quindi, a chi spende 100 dà 100, come è stato per tutti i terremoti che hanno colpito l'Italia nei decenni passati, quando lo Stato ha reintegrato le spese per intero.

ma se tutti fanno domanda, i sei miliardi sono assolutamente insufficienti, perché la coperta è corta. Capisco la contraddizione di un Parlamento e di un Governo che a sette mesi dal terremoto non sono ancora in grado di rispondere davanti ai cittadini e alle imprese un semplicissimo quesito: caro Stato, che cosa mi dai per ricostruire la mia casa?. Nessuno oggi è in grado di dirlo. Fra le altre cose, ci sono anche delle incongruenze giuridiche (lo dico ai colleghi avvocati e magistrati), perché nella norma primaria

nei provvedimenti del dottor Befera questo credito d'imposta viene ceduto alle banche e sarebbero queste ultime che sconterebbero integralmente la rata fatta di capitali e di interessi. Mi hanno già segnalato che probabilmente le banche che hanno molti dipendenti ed una struttura articolata possono avere credito d'imposta per far fronte e compensare, le piccole banche che hanno pochi dipendenti non potranno compensare. Quindi, non si capisce bene chi va ad accendere i mutui può farlo nelle grandi banche o nelle piccole banche e fino a che punto i 450 milioni che sono stati messi a garanzia ogni anno potranno o no coprire queste esigenze. Attenzione: queste cose le abbiamo dette a luglio, le abbiamo dette a settembre, le abbiamo ripetute in Commissione, le abbiamo ripetute in Aula, abbiamo chiesto al Governo di emanare delle norme che chiarissero questi aspetti. Dopo sette mesi siamo ancora qua senza aver chiarito assolutamente nulla

Io sono molto più pragmatico e, prima di criticare altri modelli che hanno risolto i problemi della gente, volevo vedere cosa combinava il nuovo modello: il nuovo modello finora non ha combinato assolutamente nulla.

cioè come un orientamento, una tendenza a ristorare integralmente chi ha avuto la sfortuna di avere la casa colpita dal terremoto. Poi il Presidente della Commissione bilancio o il Governo mi dovranno spiegare

per l'ennesima volta il campanello d'allarme sulla situazione dei territori. Dico un'ultima cosa scandalosa: stanno arrivando delle interdizioni antimafia che colpiscono non la mafia, non la 'ndrangheta, non la camorra, ma le aziende modenesi, le aziende che hanno sede nel cratere (come la Fratelli Baraldi), con i titolari di Modena, le maestranze di Modena, attraverso una surreale, lunare interpretazione della normativa antimafia, non sulla non sulla base di sentenze passate in giudicato o di procedimenti penali. Assolutamente no! Adesso non ho il tempo di leggervi (ma vi consiglio di farlo) tutte le elucubrazioni surreali secondo le quali non ci vogliono indizi, non ci vogliono prove, non ci vogliono procedimenti penali:

che non c'entrano - ripeto - assolutamente nulla con la mafia. Quindi, è un ulteriore aggravamento della situazione e lo Stato, invece di concorrere a risolvere il problema, concorre a complicarlo. I colleghi sappiano che questa interdizione deriva dal fatto che un collaboratore professionista di questa ditta, che collabora ancora con questa ditta, quattro anni fa a Bologna, come libero professionista, è stato il direttore del cantiere di un'azienda calabrese. Nell'informativa, Nell'informativa, totalmente sbagliata, lo hanno presentato come consigliere delegato di questa azienda calabrese, ma lui non era assolutamente nulla se non, per procura notarile, una persona che ha fatto il capo cantiere. il capo cantiere. Pertanto, un'azienda con 200 dipendenti, 500 dell'indotto, un giro d'affari di milioni e milioni sulla ricostruzione viene interdetta e non può più lavorare perché c'è questo collegamento, ossia perché un libero professionista che collabora con loro quattro anni fa è stato direttore dei lavori in un'azienda che lavorava a Bologna. Poiché, come dice il provvedimento, non c'è bisogno, né di prove né di procedimenti penali né di indizi, ma basta soltanto il *fumus* di un probabile pericolo che, a seguito di questa situazione, la malavita possa infiltrare aziende di persone nate a Modena, cresciute organizzate a Modena, conosciute e stimate da tutti, il risultato è che la guerra si fa alle persone oneste e perbene sul territorio, che rischiano di mandare a casa 200 dipendenti, tutti della zona del terremoto, e di mettere in crisi decine di aziende artigiane, anch'esse delle aree colpite dal terremoto, con una interpretazione vergognosa delle norme. Le norme servono per combattere la mafia, la 'ndrangheta e la camorra, non per mettere in difficoltà le aziende perbene! Altrimenti andiamo ad una eterogenesi dei fini...

apre una nuova finestra"), *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo

prosecuzione delle attività inerenti la gestione commissariale, senza quindi che possa verificarsi un qualsiasi pregiudizio delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente; in via generale, si osserva, poi, che la copertura finanziaria del provvedimento non sembra del tutto conforme alle regole contenute nella legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto riguarda gli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.6, 1.0.100, 1.0.1000, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 2.0.15, 2.0.16, 2.0,17, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.2 e 2.1. Su tutti i restanti emendamenti, il parere è di nulla osta». con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale

2.0.19 (testo 2), trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta». conformemente a quanto stabilito dalla Commissione in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.2,

delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, rendendone praticabile l'attuale dinamica che negli ultimi anni il nostro Paese ha visto crescere in maniera esponenziale e raggiungere i livelli richiesti dalla normativa

il parere del Governo è conforme a quello del relatore,

*relatore*. Signor Presidente, come ho detto nella mia relazione introduttiva, la Commissione si è a lungo interrogata sull'attuale congruenza della cosiddetta TARES e sulle dinamiche di corresponsione al criterio di tariffa piuttosto che non a quello di imposta.

Differendo, quindi, l'esazione della prima rata della TARES a luglio piuttosto che ad aprile, come previsto dalla norma, diamo la possibilità a quello che sarà il nuovo Governo di poter intervenire sulla materia riconducendo la TARES alla sua natura di tariffa, estrapolando quindi dall'imposizione TARES tutta la parte impropria Grazie, e obbligo del cittadino a pagarlo. Soprattutto quello che la Commissione auspica - come ho detto anche nella relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva svolta sul tema dei rifiuti - è che questa tariffa venga determinata con criteri Grazie, gestione degli stessi, e non già in termini di consistenza patrimoniale o di presupposte consistenze familiari che magari

una proroga dell'entrata in vigore della TARES. Abbiamo sempre sostenuto che il modo con cui il Governo ha voluto introdurre la TARES fosse un pasticcio un pasticcio per le politiche concrete di gestione dei rifiuti che si devono mettere in campo nei Comuni italiani. Si tratta di un pasticcio perché, nei fatti, si impone un ulteriore

Peraltro, colgo l'occasione per ricordare al Governo e ai colleghi della 5a Commissione che si è provato, in occasione del decreto che ha introdotto la TARES, a modificare almeno quelle parti dell'emendamento governativo che impedivano di continuare le *best practice* in alcuni Comuni in cui esse erano già in atto. Bisogna infatti ricordare che nel nostro Paese esistono numerose esperienze positive con la tariffa già in vigore, che si stava già operando nella direzione giusta. Con l'intervento della TARES si è fatto un passo indietro. Questo è il motivo per cui sarebbe stato utile prevedere una proroga dell'entrata in vigore di detta tassa. Prendo atto

Quindi, addiveniamo a questa proposta. Ci rendiamo conto che l'ultimo testo proposto dal relatore potrà comportare un qualche problema di cassa

un motivo in più per premere sul prossimo Governo affinché risolva finalmente questa vicenda, distinguendo esattamente gli oneri che bisogna pagare per gestire in maniera

mandare avanti i sindaci con questo nuovo balzello mascherato da tassa sui rifiuti, tassa che poi gli stessi sindaci sono obbligati ad imporre ai propri cittadini

In qualche modo ci adeguiamo alla ulteriore formulazione nella speranza che, nei primi mesi di attività, il prossimo Governo possa mettere mano a questa nuova tassa

di capire in modo diretto e chiaro l'efficienza del servizio fornito alla cittadinanza. Il fatto di tornare ad un concetto di tassa, scollegandolo dal pagamento di una fornitura di servizi, e addirittura di aver aggiunto da un minimo di 30 centesimi ad un massimo di 40 centesimi al metro quadrato per i cosiddetti servizi indivisibili, riducendo i trasferimenti dallo Stato centrale (che arrivano dalla fiscalità generale e che quindi sono per loro natura più equi rispetto ad un'impostazione di tipo patrimoniale), è un elemento oggettivamente molto critico che ci auguriamo possa essere modificato

esistano i requisiti, previsti esplicitamente nell'articolo 2, di condizioni di emergenza ambientale e di straordinaria necessità ed urgenza.

approfondire il tema del terremoto. La situazione, per fortuna, non è negativa come è stata presentata: ci sono molte luci nello sforzo di accompagnare l'emergenza e la ricostruzione. Resta il fatto che ci sono delle criticità pesanti, soprattutto con riferimento alla messa alla messa a regime delle procedure e all'utilizzo di criteri un po' più flessibili ed elastici per poter corrispondere meglio alle aspettative legittime dei cittadini, delle persone. In particolare, si sostiene la

va proprio in questa direzione: rispetta i vincoli di compatibilità del fondo messo a disposizione, introducendo però il principio di flessibilità,

In questa maniera si introduce il principio della flessibilità, si da cioè la possibilità di corrispondere a quella esigenza rimanendo all'interno dei vincoli di compatibilità che non possiamo non considerare. non considerare. Sono consapevole che forse in questo modo non risolviamo tutti i problemi. Però facciamo fare un passo in avanti e forse creiamo le premesse perché i commissari, esercitando la loro responsabilità e interloquendo con i territori, possano almeno parzialmente andare nella direzione che tutti auspichiamo, cioè che ci sia una copertura pari al 100 per cento dei fabbisogni di chi deve almeno ricostruire la sua prima casa di abitazione. Quindi invito e auspico che ci sia la condivisione da parte del Governo, come c'è stata dalla Commissione. Mi auguro che il presidente Azzollini, parlando della competenza della 5a Commissione, possa dare un via libera a questo emendamento. Non è forse risolutivo di tutto, ma lo è di una parte consistente di problemi.

credo che sarebbe un bel modo, almeno per me, per il mio territorio a cui faccio riferimento di chiudere un'esperienza.

ci sono molte ombre Governo-Parlamento-commissario straordinario e molte luci perché c'è stata una mobilitazione straordinaria delle popolazioni, degli imprenditori, delle maestranze, degli amministratori locali che hanno saputo spendere le somme per l'emergenza. Buio completo per quanto riguarda la ricostruzione. Ma, poiché ho visto dai banchi della sinistra anche qualche smorfia rispetto ai ragionamenti che facevo prima su un ostacolo che, invece di agevolare la ricostruzione,

che nel procedimento amministrativo cautelare antimafia viene riconosciuta all'autorità prefettizia l'esercizio di un potere discrezionale fondato sulla preliminare valutazione degli elementi di cognizione complessivamente raccolti a seguito dell'istruttoria non aventi necessariamente carattere di prova; rilevato infatti, che la normativa antimafia prescinde dall'accertamento di responsabilità penali, attribuendo significato a profili indiziari, ovvero ad eventi ipotizzati come possibili, che consentono di desumere ragionevoli legami o condizionamenti anche in presenza di coinvolgimenti non diretti nell'organizzazione criminale ma basati su fenomeni familiari o economici (...). Quindi il pericolo di infiltrazione viene basato non su prove, prove, vicende giudiziarie, avvisi di garanzia, reati commessi, ma «attribuendo significato a profili indiziari, ovvero ad eventi ipotizzati come possibili»; come nel caso di un modenese che quattro anni fa ha lavorato in un'azienda come direttore dei lavori che poi ha avuto delle disavventure giudiziarie: ecco il collegamento fra questa impresa e il pericolo che la mafia si infiltri. Informo i colleghi che tutte le cooperative rosse, i giganti della cooperazione rossa... Lasciatemi finire. Se andate a prendere le relazioni antimafia, vedete tutte le disavventure che sono capitate a questi colossi quando hanno lavorato al Sud, anche con funzionari arrestati, eccetera; non ebbene, se si dovesse applicare la *white list* con questi presupposti che ho letto, nessuno di questi potrebbe lavorare:

e queste discrezionalità non vengono applicate (il che sarebbe ancora peggio). Però, non credo che questa sia civiltà giuridica. La domanda successiva è la seguente. Quando voi avete fatto fallire un'azienda, che ha già registrato 100 milioni di euro di danni, e le maestranze rimangono a casa,

Ripeto, imprese di persone nate, cresciute, vissute e conosciute a Modena. Se andate a prendere i giornali del dopo terremoto, noterete che questa impresa è stata la prima ad intervenire all'Aquila e ad aiutare a togliere le macerie nell'emergenza, perché compie anche atti di generosità. signor Presidente, non capisco... Credo che stiamo parlando di cose molto serie, forse è stato un collega siciliano, che avrà una mentalità diversa da quella dei modenesi e degli emiliani. Noi la mafia non sappiamo cosa sia e non vogliamo saperlo, però sappiamo che ci sono le persone oneste e non vogliamo che lo Stato venga da noi non ad aiutarci per la ricostruzione, ma ad intralciare

Nel 2010, in Italia, la spesa nazionale per la gestione dei rifiuti, delle acque reflue e delle risorse idriche aveva un'incidenza sul PIL del 2,2 cento della spesa proveniva dal servizio di gestione dei rifiuti, settore per il quale rimaniamo ancorati al binomio discarica-incenerimento. Sono stati però gli investimenti dei produttori specializzati privati, ossia di quelle imprese che hanno per attività principale la produzione di servizi ambientali per la vendita a terzi, a far registrare la quota maggiore sul totale della spesa nazionale, a fronte di una percentuale del 2 per cento dei produttori specializzati pubblici. L'ammontare della spesa ambientale erogata dal complesso delle amministrazioni regionali italiane nel 2010 è stata corrispondente ad una spesa media di soli 71,6 euro per abitante, con un'incidenza sul prodotto interno lordo pari allo 0,28 Rispetto al 2009, la spesa è diminuita di oltre il 15 per cento. Questa quota è ulteriormente calata nel 2011 e nel 2012 per effetto della crisi. I settori ambientali cui è stata destinata la quota maggiore della spesa sono: protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie; uso e gestione delle risorse idriche; protezione della biodiversità e del paesaggio; gestione delle acque reflue; uso e gestione delle foreste. Questo è l'elenco delle cose che dovremmo fare, cui dovremmo dedicare gli investimenti, perché non di spesa a perdere, ma di investimento per il futuro si tratta. Nulla di tutto ciò è stato fatto. Si è invece colta l'occasione per qualche norma di favore, per qualche balletto elettoralistico dell'ultimo momento. La maggioranza che ha sostenuto il Governo ha ritenuto di introdurre un ulteriore balzello: la TARES. Doveva essere la novità di gennaio ma era troppo vicina alla stangata dell'IMU e soprattutto, sarebbe arrivata subito prima delle elezioni. Così - strategicamente - è stata prima rinviata ad aprile 2013 e poi, con il voto odierno della Commissione ambiente, si è pensato di spostarla al prossimo mese di luglio. Ma la sostanza non cambia perché, mentre ancora non viene restituita ai cittadini italiani l'IVA pagata sulla tariffa rifiuti, la nuova imposta - scatti essa da aprile o da luglio - comporterà comunque un ulteriore appesantimento dei tributi a carico dei contribuenti e dei proprietari di immobili, senza riguardo alcuno al reddito ed in barba ad ogni criterio di equità e progressività. Non solo essa si basa, come l'IMU, su una situazione generale dei dati catastali iniqua e opaca (in cui immobili di pregio valgono meno di alloggi popolari) ma essa viene ad assorbire anche i servizi di illuminazione e manutenzione stradale. Essendo una tariffa, dovrà coprire per intero un costo dell'amministrazione rappresentato non solo dalla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa

del disconoscimento di imposte che si sono prima convintamente votate e che improvvisamente vengono disconosciute da quegli stessi che le hanno volute ed introdotte, che si potrà risolvere un problema di equità ed equilibrio fiscale come quello che soffre il nostro Paese.

ma soprattutto potessero, essere valorizzati in impianti che, soprattutto nelle regioni del Nord, ci sono e sono efficienti ed efficaci.

questo disassamento in avanti, questa proroga della TARES che, voglio sottolinearlo ancora una volta, mi sembra assolutamente inconcepibile perché pone un ulteriore balzello su cittadini già così tartassati tassa che credo sia stata una cosa veramente scellerata, mi si conceda questo termine, che forse è anche riduttivo.

un contributo positivo, dichiara il suo voto di astensione. Signor Presidente, la accelerazione impressa alla conclusione della legislatura ha consentito, fra l'altro, ai due partiti maggiori di interdire definitivamente anche solo la prima fase dei lavori in Commissione ambiente sul disegno di legge del collega Vincenzo De Luca inerente alla rivisitazione complessiva del settore della gestione dei rifiuti. Eppure, solo la via maestra di una sistematica definizione di compiti, ruoli e livelli istituzionali potrà - per via legislativa - tentare di dare ordine a un settore dalla straordinaria valenza economica, di strategico valore sociale ed ambientale e certo espressione non ultima di una dimensione culturale del vivere e della identità di un popolo. Si tratta di un settore dove invece abbiamo a che fare con un vasto degrado, con una dilagante criminalità, con una preoccupante inerzia dei pubblici poteri. Non stupisce, quindi, che quest'ultimo - all'apparenza - atto dell'Aula del Senato repubblicano in questa legislatura sia ancora - mestamente, mi permetto di dire - un atto derogatorio di termini; né stupisce che a proporlo sia questo Governo, che anche in questo settore ha dovuto rincorrere emergenze anche - come in alcuni casi contenuti nel decreto - decisamente puntuali. La 13a Commissione ha introdotto alcuni emendamenti qualificanti, che integrano opportunamente il decreto. L'accoglimento parziale del primo di tali emendamenti implica in ogni modo una riflessione aggiuntiva sul tema TARES da parte del prossimo Governo. Il voto finale sul disegno di legge di conversione sarà favorevole, accompagnato, peraltro, dall'auspicio di un generale cambio di mentalità, di una marcata assunzione di responsabilità da parte di soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti anche in questo decreto di conversione. Ma soprattutto dall'auspicio che il Parlamento riesca, nella prossima XVII legislatura, ad intervenire in modo complessivo e sistematico sul tema dei rifiuti. Presidente, il nostro voto sarà favorevole senza alcun entusiasmo, ma piuttosto come un atto dovuto perché a Camere sciolte non si può fare altro che approvare un decreto che conteneva quelle proroghe, ma non si può da noi certo pretendere entusiasmo nel dover prorogare per un'ennesima volta le norme riguardanti l'emergenza dei rifiuti in Campania,

ad esempio, il ruolo delle Province, che è assolutamente difforme da tutto quello che succede nel resto d'Italia e che qui invece viene prorogato senza alcun cambiamento. Non possiamo avere alcun entusiasmo nell'accettare la proroga per quanto riguarda i rifiuti che hanno un alto potere calorifico e che non dovrebbero più essere smaltiti in discarica. È una proroga di di un altro anno, quando in realtà quella norma andrebbe cancellata perché non ce l'ha chiesta l'Europa; è stata frutto dell'operato del Governo Berlusconi di qualche anno fa che voleva provare a realizzare i termovalorizzatori in ogni ambito provinciale ed era una evidente forzatura ideologica che poi non ha portato a niente. Quindi non possiamo essere entusiasti di un provvedimento del genere e l'unico motivo per cui invece

in un disegno di legge che la nostra Commissione ha esaminato a lungo nei mesi scorsi e che la Camera però si è tenuta per troppo tempo (per oltre sei mesi) e ci ha restituito soltanto il giorno prima dello scioglimento delle Camere, impedendo così l'approvazione di molti provvedimenti utili per l'ambiente, per la semplificazione che sempre viene richiesta e che avrebbero potuto

Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, come in parte ha evidenziato la discussione, non è, anche per le modifiche che lo hanno riguardato, la mera proposizione di una proroga termini. alcune norme che hanno un significato politico e anche di verifica rispetto alle volontà, alle posizioni e alle coerenze delle forze politiche presenti in questo Parlamento e ha assunto, nelle modifiche apportate con alcuni emendamenti, anche un significato ulteriore rispetto ad un'espressione che oggi il Senato darà dal punto di vista politico sulla insoddisfazione, sulla inaccettabilità e sulla carenza dal punto di vista istituzionale e strutturale dell'imposta sui servizi che con questo provvedimento verrà differita. Rispetto alla prima famiglia di questioni che hanno un significato politico, nelle proroghe che sono state inserite sulle gestioni commissariali da parte del Governo in questo decreto-legge esiste quella dei rifiuti e del commissariamento relativo alla Regione Campania. Si tenga presente che i lavori parlamentari di questa legislatura si aprirono con l'emergenza Campania e questo è il quarto o il quinto provvedimento con il quale si proroga la situazione emergenziale.

il commissariamento che oggi è prorogato veniva presentato dal Governo Berlusconi, dicevano che non era necessario un provvedimento commissariale, che non erano necessarie norme straordinarie e che hanno votato contro tutte le proroghe di cui quella di oggi è la buona ultima. Come a dire che a seconda di chi siede nei banchi del Governo i problemi e i provvedimenti hanno un significato tutt'affatto diverso. come il commissariamento e le norme straordinarie relative alla gestione dei rifiuti in Campania sono state volute da questa parte politica, con coerenza oggi votiamo quella parte del provvedimento che prevede la proroga la proroga di quelle norme volute dal Governo Berlusconi e che hanno, nella grande emergenza nazionale che ha riguardato la gestione dei rifiuti in Campania, certamente portato lentamente ma inesorabilmente ad una soluzione positiva. Il provvedimento ha poi acquisito una nuova importanza con gli emendamenti presentati dalla Commissione e da diversi colleghi che sono intervenuti qui in Aula (per il Gruppo del PdL il senatore Giovanardi) per portare ragionevolezza ed equità rispetto al processo di indennizzo per i danni ai terremotati, per consentire che queste risorse vengano innanzitutto spese e quindi siano un sollievo concreto ed anche, dal punto di vista economico, un'occasione di sviluppo legata comunque alla ricostruzione, che certamente di doverosità morale verso chi ha subito dei danni gravissimi in un cataclisma naturale, ma con la ripresa delle attività, con la destinazione di fondi, con la ricostruzione è anche, in questi momenti, una

Anche su questo il Governo ha stabilito delle chiusure. Rimane comunque l'opportunità che gli indennizzi diventino più equi e i miliardi di euro già accantonati possano essere spesi

non strangolato da una legge di stabilità e da un voto di fiducia, rispetto all'ingiustizia legata alla TARES. Questa tassa sui servizi aumenta del 30 per cento indiscriminatamente, senza che i Comuni lo possano modificare, il costo delle tariffe dei rifiuti che sono vigenti, e snatura - com'è stato ricordato - la stessa logica della tariffa ambientale e del principio del diritto ambientale per cui chi base alla quale quindi ciascuno dovrebbe corrispondere un contributo in funzione dei rifiuti che produce. Questo rappresenta il modo in cui nell'ultima legge di stabilità si è travisato un impianto normativo previsto nei decreti di federalismo fiscale e che prevedeva sì una tassa sui servizi generali ma non come una sovrattassa o come un'addizionale o come un automatismo, quindi prescindendo dai servizi e da chi

ai proprietari di prima casa, che sono stati sottoposti in maniera inusitata all'IMU, verrà richiesta anche un'ulteriore tassa sui servizi che colpirà lo stesso bene

che in questo regime di tassazione degli ultimi mesi, che colpisce dei beni fondamentali come la prima abitazione e aggiunge, senza neanche la possibilità per i Comuni di poterle modificare, delle sovrattasse facendole pesare sulle famiglie in questo momento di crisi, ci sia

Il senatore Ferrante nella sua dichiarazione di voto ha espresso la mancanza di entusiasmo, pur mantenendo invece il voto a favore su questo

di serietà con quell'esercizio. Ma non credo che chi ha a cuore lo Stato di diritto - e un radicale è uno di questi - possa votare a favore di un provvedimento che ha un articolo che inizia in questo modo: deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo (...)». L'Italia è fondata sulla deroga dello Stato di diritto e la creazione di un commissario per qualsiasi cosa. Non si è riusciti in cinque anni, malgrado i commissariamenti (e sono migliaia i commissari in Italia), a gestire una emergenza che sia una. Questa legislatura si conclude ancora una volta con la conferma di una classe dirigente che, proprio perché non rispetta la propria Costituzione, non può far applicare nessuna legge. Quindi ci asterremo.

purtroppo è la stessa disattenzione con cui alla Commissione di vigilanza RAI - e mi dispiace che non ci sia in Aula il presidente Zavoli - si è ulteriormente calpestato lo Stato di diritto in Italia, conferendo all'Ufficio di Presidenza la gestione delle fasi finali di questa campagna elettorale,

Si stanno prendendo delle decisioni senza sapere neanche quante saranno le coalizioni che parteciperanno alle elezioni né quante saranno le liste all'interno delle coalizioni stesse. a una RAI, che è in drammatico calo di ascolto, dei minuti che non si sa a quante persone andranno distribuiti e si lasciano andare sempre i soliti all'interno di trasmissioni di intrattenimento e di approfondimento che sono al di fuori di qualsiasi tipo di regola.

mi si dice di sì. Spero però che non si vada a peggiorare ulteriormente, perché tutte le volte che la si riconvoca, finisce così, la questione. Siccome il presidente Zavoli sarà ricandidato nella prossima legislatura, gli auguro di fare altro per i prossimi cinque anni.

onorevoli colleghi, questo sarà il mio ultimo intervento in quest'Aula (sottolineo in quest'Aula, perché continuerò dall'esterno, in modo libero e assolutamente indipendente, a condurre tutte le mie battaglie politiche

Intervengo per esprimere la mia delusione, rafforzata da questa breve esperienza in questo Senato della Repubblica, per l'insensibilità dimostrata dal Governo ormai defunto. Insensibilità rispetto a quanto sta succedendo nel mondo esterno, dal quale coloro che rappresentano questo Parlamento evidentemente sono molto lontani, e da molti anni. Insensibilità anche nel dare delle risposte alle interrogazioni che la sottoscritta aveva presentato in questi brevi due mesi di impegno all'interno del Parlamento.

Nessuno ha preso posizione in merito a questa interrogazione. Me ne dispiaccio perché, da ex malata di cancro, posso capire che, con la situazione economica che vivono

Voglio anche citare un argomento che mi sta molto a cuore. Mentre noi sostenevamo un Governo tecnico, l'assenza della politica ha generato preoccupanti azioni da parte di enti che si sono presi la libertà di emanare

Il 2013 si apre quindi all'insegna di una novità per gli invalidi civili al 100 per cento titolari di una pensione di invalidità. Si tratta di una prestazione economica erogata a favore dei lavoratori per i quali non è stata accertata la completa e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità fisica e mentale. Chiedo che si assumano provvedimenti, perché l'assenza della politica ha lasciato spazio ad interventi assolutamente non etici.

grazie ad una disponibilità, di portare avanti le nostre questioni. Non sono andate in porto quelle sulla legge elettorale e sulla riforma costituzionale, ma non perché non ve ne fosse la disponibilità, perché in Commissione

Grazie, signor Presidente. i colleghi abbiano apprezzato il contributo, che peraltro è importante, non solo suo, ma dei Gruppi che rappresentano le minoranze linguistiche e che concorrono ad assicurare il pluralismo democratico del nostro Paese. Colgo di nuovo l'occasione